che da parte della maggioranza, della Lega ma in realtà anche di tutto il centrodestra, ci sia la volontà di affrontare questo problema. Certo che dobbiamo dare dignità a questi lavori; certo che la remunerazione deve corrispondere ad una reale esigenza del lavoratore e non deve essere sfruttamento, ma deve essere dignitosa. Si tratta di capire come arrivare a questo obiettivo. Noi abbiamo semplicemente ribadito che per noi il salario minimo stabilito

che il parametro che la direttiva europea mette in evidenza come obbligo, intimazione ad andare verso la tutela o comunque verso una legge che tutela il salario minimo è che

i rischi di cui parlavamo sono legati al fatto che col salario minimo stabilito per legge c'è il rischio di appiattimento verso il basso dei salari mediani (questo è un rischio reale), di depotenziamento della contrattazione collettiva e delle varie tutele, anche significative, che sono state introdotte anche grazie alla contrattazione collettiva di secondo livello.

Per queste ragioni, intendiamo ribadire che vogliamo superare la criticità e risolvere questo problema, perché ovviamente c'è grande attenzione a quei

anche, come ha fatto questo Governo di centrodestra, affidare al CNEL il discorso di un piano d'azione, proprio per rafforzare la contrattazione collettiva di secondo livello. Questo è quello che vogliamo fare noi. Non puntiamo sul salario minimo per legge, ma sui minimi salariali contrattuali esigibili, attraverso il rafforzamento e il potenziamento della contrattazione collettiva.

quello che propone l'opposizione, ma altrettanto deve essere rispettabile quello che propone la maggioranza. Ricordo, peraltro, che come Lega abbiamo presentato un progetto di legge che va proprio nella direzione del rafforzamento della contrattazione di secondo livello, nel quale si vuole intervenire sui trattamenti economici accessori, tenendo conto anche del parametro legato al costo della vita e alla produttività, che non significa tornare alle vecchie gabbie salariali, che era un sistema rigido, ma prendere atto di una realtà che qualcuno non vuole vedere, ossia che nelle grandi città la vita costa molto più che nelle periferie e che ci sono alcune zone del Paese dove la vita costa di più rispetto ad altre zone del Paese. Non vedere questo significa essere completamente scollegati dalla realtà.

quindi, è una delle strade che possiamo intraprendere ed è quello che chiediamo noi come Lega, che abbiamo ribadito nel nostro disegno di legge, proprio perché vogliamo risolvere il problema rafforzando la contrattazione collettiva di secondo livello, quindi senza intervenire

la serietà dell'intervento del senatore Romeo, che non condivido nel merito ma sicuramente nel metodo, meriti una risposta, che mi auguro possa essere considerata altrettanto seria, anche se probabilmente non condivisa. È evidente che il problema dei lavoratori poveri che non riescono ad arrivare non a fine mese, ma neanche a metà del mese, è un problema reale e concreto che mi sembra evidente

lavora al di sotto dei nove euro lordi l'ora, è evidente che la protezione del contratto collettivo nazionale non è sufficiente per dare dignità allo stipendio, al lavoro. Affermare che soltanto attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva si può raggiungere l'obiettivo, sta nei fatti e nei dati che non sia così. secondo luogo, parlare di contrattazione di secondo livello e di trattamento economico complessivo può avere un senso, ma non dobbiamo dimenticare che la gente va a fare la spesa con il netto in busta paga e non con il trattamento economico complessivo. Quindi, quello che arriva al netto in conto corrente è quello che io posso usare per vivere. Tutto il resto serve, ma non risolve i problemi emergenti di chi oggi non arriva alla terza settimana. Non vi è alcun rischio di depotenziamento della contrattazione collettiva e del ruolo delle forze sindacali nel momento in cui si approva una norma che prevede un limite minimo legale orario. orario. Nello stesso momento in cui io fisso il principio che deve essere la norma ad indicare il salario minimo orario legale, rafforzo anche la contrattazione collettiva, perché le nostre proposte, quelle delle opposizioni, totalmente unite su questo fronte, vanno a rafforzare anche la contrattazione collettiva. metto al centro la contrattazione collettiva e la protezione che quella contrattazione dà ai lavoratori. Dall'altra, dico che però quella contrattazione non può partire da un livello salariale che sia inferiore alla cifra indicata di nove euro l'ora. Signor Presidente, concludo paventando un rischio. In questa fase abbiamo visto un forte allentamento delle politiche di assistenza al reddito per chi perde il lavoro, per chi il lavoro non riesce ad averlo, per chi esce dal mondo del lavoro. Aver eliminato un sistema universale di accompagnamento al reddito (non cito il reddito di cittadinanza, ma parlo di uno strumento universale di assistenza e di accompagnamento a chi non ha un lavoro) rischia di portare una fascia sempre più debole della popolazione ad accettare lavori che non hanno dignità salariale. E questo è un altro effetto collaterale delle politiche che questo Governo sta attuando. *(Applausi)*.

Signor Presidente, accetto la sollecitazione del capogruppo Patuanelli per parlare di un tema veramente delicato. Se ognuno di noi avesse la soluzione ideale e perfetta, sarebbe un'utopia e, francamente, nessuno di noi pensa che quello che dice l'altro sia completamente sbagliato e che chi invece sostiene diversamente abbia

(che vuol dire 6,50 euro netti, molto meno di quanto molti contratti di contrattazione collettiva prevedono per i propri lavoratori), in in realtà, invece di favorire la minoranza che ha dei contratti capestro, danneggerebbero la maggioranza che invece ha dei contratti migliori. Il rischio, allora, è che quel tipo di previsione legislativa, invece di favorire un miglioramento della vita

è vero, ma riguarda categorie che fino a ieri ne erano esenti: insegnanti, infermieri, autisti di autobus, cioè persone che hanno una contrattazione collettiva e che guadagnano in teoria uno stipendio che un tempo si sarebbe definito normale. Oggi, a causa dell'inflazione e a causa del fatto che i salari non sono stati adeguatamente incentivati in questi anni, vengono considerati i nuovi poveri. E allora, sempre per fare un ragionamento e per fare delle proposte, noi per esempio abbiamo presentato una proposta di legge che prevede che il lavoratore partecipi agli utili di impresa.

e quello che una volta si chiamava padronato si crei un rapporto di leale collaborazione reciproca, in modo tale che tutti si sentano parte di una squadra, per il bene dell'azienda e per la qualità. Ma soprattutto, dove questo avviene (per esempio in Germania), ci sono stati degli elementi di crescita economica delle aziende che lo applicano che sicuramente mancano in questa fase nel nostro Paese. Se il tema è quel pezzo di lavoratori fragili o fragilissimi che in questo momento hanno dei contratti capestro, non è indebolendo la contrattazione collettiva

tuttavia che le due cose cozzino insieme, perché, se io sono libera di contrattare, non devo avere un *incipit* iniziale. E soprattutto, non avendo quell'*incipit* iniziale, posso andare molto più avanti e molto oltre rispetto ai 9 euro lordi, che sono più o meno 6,50 euro netti e che non sono concepibili nella stragrande parte dei contratti. Ciò vorrebbe dire che si dà l'autorizzazione, a quelli che guadagnano di più, di guadagnare di meno. Bisogna tutelare i fragili, anche dando delle multe salatissime alle multinazionali che sfruttano i lavoratori. Facciamo allora adeguate politiche di controllo, grazie ai sindacati. Ma, visto che la contrazione collettiva e il ruolo del sindacato sono centrali nella nostra Costituzione, delle non è che si può salvaguardare la Costituzione quando ci fa comodo e, quando invece va contro i nostri ideali, diciamo che vale ma quanto basta. sindacati e la contrattazione collettiva sono stabiliti in Costituzione e la sentenza dell'Unione europea non dice che è obbligatorio il salario minimo, ma dice che, dove dove non c'è la contrattazione, bisogna corrispondere il salario minimo, perché le due cose sono antitetiche.

l'idea che un salario minimo faccia rivedere al ribasso le contrattazioni sugli altri redditi e sugli contrastato dalla realtà dei fatti. In Germania, dove esiste il salario minimo, la contrattazione collettiva ha portato al 31 per cento in più di crescita dei salari, in Italia siamo scesi del 2,9 per cento. i contratti non vengono adeguati e l'abbiamo ripetuto tutti, proprio perché la contrattazione collettiva va rafforzata, cosa che il nostro emendamento sull'introduzione del salario minimo prevedeva, perché è la contrattazione collettiva veramente rappresentativa che deve essere sostenuta. Infine, noi sentiamo raccontare dalla maggioranza di questa crescita strepitosa dell'occupazione. Ricordo che è un *trend* in vigore dal 2021, quindi ben venga la crescita. Peccato che il PIL sia ritornato a cifre da prefisso telefonico dello zero virgola e questo dimostra che alla crescita dell'occupazione corrispondono salari poveri, altrimenti il PIL crescerebbe. Quindi la realtà dei fatti smaschera il vostro finto interessamento alla tutela dei lavoratori poveri. State dando l'ennesimo schiaffo a tre milioni di lavoratori poveri.

possibilità e dell'efficacia della contrattazione di secondo livello, che non è una novità perché, insisto, il modello su due livelli vale dal 1993, quindi abbiamo alle spalle una discreta esperienza. La seconda ragione per cui abbiamo bisogno di un salario minimo e di fissare una cifra sotto la quale non andare

anzi, il salario minimo rafforzerebbe la contrattazione, innalzando la base da cui partono i salari.

rinnovato i contratti della scuola e previsto 7 miliardi per i rinnovi dei contratti di tutto il pubblico impiego, quindi di cosa state parlando?

vorrei evitare di fare *bagarre* su una cosa che riguarda moltissimi lavoratori e lavoratrici.

che non si può andare sotto e quando uno fa l'appalto deve sapere che appalta. Anche la pubblica amministrazione, quando appalta un servizio, deve sapere che lo deve dare, se c'è un rispetto dal punto vista economico e contrattuale. Ci sono

cento della contrattazione collettiva di questo Paese, cioè il 97 per cento dei lavoratori coperti da contrattazione collettiva, porta la firma almeno di CGIL, CISL e UIL, oltre che di altre sigle. Quindi attenzione, quando si citano i numeri.

semplice, che meriterebbe qualcosa di più rispetto al teatrino della politica politicante, che troppo spesso viene tirata in ballo su vicende come queste che intende lucrare al mercato della facile politica e della raccolta del consenso spicciolo su questioni che meriterebbero un approfondimento ben più consistente e anche una coerenza di fondo. fondo. A me fa piacere - o, meglio, per certi aspetti sorprende - sentire in quest'Aula alcune affermazioni da parte di colleghi che, quando svolgevano funzioni di rappresentanza di significativa importanza, la pensavano in maniera diametralmente opposta. La collega senatrice Camusso si è alzata ora magnificando le magnifiche e progressive sorti del salario minimo. se sia la stessa segretaria generale della CGIL che, a suo tempo, incontrando i rappresentanti del Governo dell'epoca, significativamente di centrosinistra, diceva testualmente che l'introduzione del salario minimo avrebbe la funzione di «indebolire la contrattazione collettiva» e «creare le condizioni per un futuro di povertà diffusa». La senatrice Camusso, all'epoca segretario generale della CGIL, diceva una cosa giusta: «non «non c'è alcuna ragione al mondo che giustifichi l'intervento del Governo sulle regole contrattuali». Ora si dà il caso che il Governo dell'epoca avesse un torto, probabilmente, quello di essere riformista e di centrosinistra, che quindi, per una concezione massimalista, non doveva essere in alcun modo agevolato, ma in tutti i modi contrastato. Peraltro, anche chi è venuto dopo di lei alla guida del più importante sindacato italiano (mi riferisco a Maurizio Landini) nel 2019 sosteneva a chiare lettere, testualmente: «sono le parti sociali (a fare il salario minimo), quando rinnovano i contratti nazionali». È esattamente quello che sosteniamo anche noi.

del salario minimo indebolisce i lavoratori, non li rafforza». Anno di grazia del Signore 2021, ministro del lavoro Andrea Orlando.

nei due minuti che mi sono concessi, visto che già ieri siamo intervenuti su questo tema, mi premeva dire due cose, una per il suo tramite al senatore Romeo, che probabilmente confonde la defiscalizzazione e il cuneo fiscale con i rinnovi dei contratti collettivi. *(Applausi)*. Visto che parla di cose che, a mio avviso, conosce un po' per sentito dire, forse è il caso di riportare un po' di verità su questo tema. Allo stesso modo, se abbiamo più di 800 contratti collettivi nazionali registrati e oltre 3 milioni di italiani che stanno sotto la soglia dei 9 euro,

presentato un disegno di legge che affronta il tema. Ritorno allora a quanto detto ieri: siccome la direttiva non obbliga a scegliere tra la contrattazione collettiva e la legge, ma vi dice che contrasta il lavoro povero, è evidente che abbiamo bisogno di una soglia sotto la quale non si può andare. Non me ne vogliano i colleghi quando dicono che questo indebolisce la rappresentanza sindacale o la contrattazione collettiva, perché se a dirlo sono state la Banca d'Italia e la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nell'ultima settimana, evidentemente il tema è che il problema dei salari in Italia esiste, eccome.

facoltà per due minuti, perché avremmo esaurito i tempi.

portato a una soluzione. Si vuole continuare a non affrontare un problema che tiene bloccato l'intero comparto di un Paese

per valutare il fatto che non ci fossero risorse scarse e quindi venisse meno il presupposto per le gare e le procedure di evidenza pubblica. lettera di messa in mora della Commissione, che non basterà il lavoro del tavolo tecnico e della mappatura. Pertanto, in questo emendamento vi chiediamo semplicemente di applicare la normativa europea e la direttiva servizi per chiedere il ricorso alle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra l'altro, questo emendamento tiene in equilibrio il riconoscimento degli investimenti effettuati agli attuali titolari di strutture, quindi indennizza i concessionari uscenti e definisce tutele occupazionali,

disegno di legge di delegazione europea costituisce uno dei momenti più importanti di partecipazione dell'Italia agli adempimenti degli obblighi dell'Unione europea. Come sappiamo bene, purtroppo, l'Italia non si è sempre contraddistinta per l'adeguamento agli obblighi comunitari, sia per un tema di vischiosità dell'ordinamento nazionale frammentato tra lo Stato e le Regioni, sia, più in generale, per una tendenza sbagliata del nostro Paese ad assumere obblighi normativi vincolanti nell'ordinamento.

Credo che possa riprendere, una ventina su temi importanti, dalla *cybersecurity* alla tutela dei lavoratori esposti a elementi cancerogeni, come l'amianto ed altri, quindi sono tutti provvedimenti importanti. Tra questi ricordo un emendamento di cui ieri abbiamo discusso a lungo, presentato dal collega Costa alla Camera, che è diventato oggetto di ampia discussione all'interno del presente disegno di legge, che si collega alla normativa europea sul principio di non colpevolezza. Non posso non rimarcare che ci sono state occasioni mancate in questa discussione, a partire da quella che citavo prima sulle concessioni balneari, su cui continuiamo a rimanere ostaggio di una parte della maggioranza, che fatica a enunciare un principio molto semplice, che si chiama libera concorrenza.

la proposta sul salario minimo, ma anche rispetto a un tema che riguarda oltre tre milioni di italiani e che da Bankitalia alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ci viene posto come rilevante per il Paese, cioè quello dei salari bassi e del lavoro povero. Non avete ascoltato alcune delle nostre richieste, ma confido sia nel sottosegretario Siracusano sia nel ministro Fitto un suggerimento di metodo venga raccolto, cioè che, quando si lavora sulla legge di delegazione europea e si devono indicare quali procedure di infrazione chiudere per prime, la scelta non dipenda da valutazioni politiche del Governo,

Quando si adottano leggi che delegano il Governo a chiudere procedure di infrazione, la logica dovrebbe essere quella di partire prima da quelle che hanno già una sentenza di doppia condanna

non perché ci siano parlamentari che non vogliano lavorare di giorno o di notte, in qualsiasi orario, ma perché svolgere una discussione con il favore delle tenebre come ieri notte anziché con il favore della luce del giorno non è degno di uno dei temi più delicati che riguardano il rapporto tra l'Italia e l'Unione europea e questo problema - mi ripeterò rispetto a quanto detto nel mio intervento in discussione generale generale - non si risolve solo con uno strumento tecnico-giuridico, che oggi è quello della legge di delegazione europea e poi sarà quello della legge europea, perché è culturale: significa identificare e accorciare la distanza che passa tra la fase ascendente, in cui si assumono obblighi

che agli obblighi europei si possa adempiere o no a seconda del colore politico del Governo. Questo è l'errore di fondo per il quale l'Italia non riesce a essere in linea con gli obblighi europei. Azione saremo sempre favorevoli tutte le volte in cui l'Italia si conformerà a obblighi che ha già assunto - ed è il motivo per il quale dichiaro il voto favorevole alla legge di delegazione europea - ma mi raccomando: raccogliete gli *input* e gli stimoli che vi stiamo dando come opposizione, perché su questo si fonda la credibilità del nostro Paese quando assume obblighi vincolanti non solo a livello europeo, ma anche interno e nazionale.

tra il nostro Paese e le istituzioni europee, infatti, sono contraddistinti, oggi ancor più che in passato, da proficue relazioni bilaterali. L'approccio assertivo del Governo Meloni sta producendo risultati evidenti nella gestione dei flussi migratori, ad esempio. Ricordiamo l'importanza del contributo italiano nella firma del *memorandum* d'intesa con la Tunisia, un vero e proprio simbolo del cambio di paradigma che consiste nella difesa dei confini esterni dell'Unione europea, fermando a monte i trafficanti di esseri umani. Ricordo inoltre il pagamento della quarta rata del PNRR all'Italia, che è diventata così il primo Paese in Europa a riceverla. Ebbene, l'atto che votiamo oggi è un ulteriore tassello di queste relazioni di collaborazione, pace e sicurezza con la stessa Noi siamo europeisti della prima ora, lo siamo da sempre. L'appartenenza all'Unione europea per noi è motivo di vanto. Oggi, però, è cambiato l'approccio: ci stiamo rendendo conto concretamente che si può essere in Europa a testa alta, portando avanti gli interessi della nostra Italia. Grazie a questo Governo e a questa maggioranza abbiamo ritrovato una giusta dose di protagonismo. La postura dell'Italia è sicuramente cambiata. I primi risultati li stiamo vedendo. Penso, ad esempio, alla lotta contro le carni sintetiche, tema su cui i quattordici Stati membri dell'Unione europea si sono allineati alla posizione italiana e di questa maggioranza, a tutela della qualità dei nostri prodotti e delle eccellenze del nostro *made in Italy*. Dobbiamo proseguire su questa strada e questo Governo lo sta facendo concretamente, per sconfiggere quelle ideologie *green* che non tutelano l'ambiente, così come non tutelano, ma al contrario danneggiano, i nostri imprenditori e i nostri territori.

dalla legge 24 dicembre 2012, n. 34, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Europa stessa. Il disegno della legge oggi in esame prevede, nello specifico, il recepimento di diciassette direttive e di sei regolamenti, che hanno come oggetto questioni e materie di grande rilevanza per la vita di cittadini e imprese della nostra Nazione. Vorrei soffermarmi su alcuni dei diciannove articoli presenti nel provvedimento. Ad esempio, l'articolo 3 è relativo a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza dell'Unione europea.

Questi numeri ci fanno capire quanto sia oggi importante difendere e proteggere il cyberspazio esattamente come lo spazio fisico che è attorno a noi. Il tema di cybersicurezza è dunque di fondamentale importanza per la sicurezza delle nostre istituzioni e dei nostri cittadini. Il dato, infatti, può apparire come qualcosa di freddo, ma invece appartiene alla vita di ciascuno di noi. Ecco perché è essenziale e cruciale implementare le misure a sua protezione. La direttiva in questione rafforza il livello della *cyber*-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. A proposito di lavoro, è utile citare gli articoli 8 e 9. L'articolo 8 riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Il nostro Gruppo, signor Presidente, è particolarmente sensibile a questo tema, come dimostra il fatto che, sin dall'inizio della legislatura, si è mobilitato in favore della sicurezza del lavoro e dei malati oncologici, non da ultimo, con la legge sull'oblio oncologico, recentemente approvata in via definitiva. L'articolo 9, invece, riguarda l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Come dimostrano diversi studi al riguardo, per affrontare la sfida epocale della crisi demografica, tentando di invertire la tendenza negativa, serve, sì, cambiare l'atteggiamento culturale, ma servono anche concretamente lavoro e sviluppo. Serve pertanto far crescere i tassi di partecipazione, di occupazione e di retribuzione femminili al mondo lavorativo. provvedimento, in conclusione, rafforza la sinergia dell'Italia con l'Europa. Continueremo a lavorare in tale direzione, consapevoli delle potenzialità della nostra Nazione e dell'importanza di promuovere nelle sedi europee tutte le azioni necessarie per salvaguardare gli interessi nazionali; in poche parole, per fare gli interessi dell'Italia e degli italiani. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo UDC-Coraggio Italia- Noi Moderati-MAIE.

questo atto ci dà l'occasione di fare il punto su alcune questioni che in ambito europeo sono oggetto di una discussione importante e forte e anche per fare un po' di luce su alcune strumentalizzazioni che

è in grado di fare per rafforzare il processo di unità tra gli Stati, ma anche per traghettarli verso obiettivi nuovi di modernizzazione, di ambientalizzazione

ambientale, con una forte crescita occupazionale e un miglioramento della qualità del lavoro nel nostro Paese. Parto dal tema importante della parità di genere, soprattutto per quanto riguarda i ruoli nelle società di amministrazione. Abbiamo ancora un basso di partecipazione delle donne, soprattutto per quanto riguarda i ruoli apicali, ed è ineludibile l'obiettivo di aumentarlo. Da questa Da questa questione di civiltà ne passano alcune altre grandi, che attraversano il dibattito politico. Pensate al tema del salario: è ingiustificato, ingiustificabile e gravissimo che le donne abbiano

che spesso avviene nelle case. *(Applausi)*. Noi affrontiamo il dibattito sulla violenza e sulle storture nelle vite familiari solo dall'angolatura del tema culturale, che è sacrosanto e che ovviamente deve vederci tutti impegnati, a partire dalla scuola, dalla società e dai messaggi che lanciamo. Non ci fermiamo a riflettere però su una delle condizioni fondamentali affinché le donne abbiano una loro autonomia, cioè la loro indipendenza economica *(Applausi)* e il fatto di far valere il loro lavoro, il loro ingegno e il loro talento tanto quanto gli uomini

che, a differenza di altri Gruppi, considero il fatto di avere una Presidente del Consiglio donna un valore per tutte noi. *(Applausi)*. La penso in maniera diametralmente opposta a Giorgia Meloni su molte questioni, ma non possiamo non riconoscere che questo sia un obiettivo di avanzamento della politica e della società, a cui ne deve corrispondere però uno importante

L'altra questione - e poi vengo ai due temi più spinosi - è quella del rafforzamento nelle nostre imprese, ma anche nella pubblica amministrazione, di tutte le attività che devono servire alla cybersicurezza. Mi scuso tantissimo con i colleghi di Forza Italia, se parlo di cybersicurezza e di donne. Capisco che la discussione sarà sicuramente più interessante, però vi pregherei, almeno su questo, di fare un minimo di attenzione. Le nostre imprese hanno un problema di modernizzazione riferito a questo e i dati sono impressionanti. Ancora ieri c'è stato un caso

di cybersicurezza *(Applausi)* che ha dato una struttura, una rete, sulla base della quale poi lavorare con le singole attività delle singole imprese. Purtroppo, però, il *deficit* di competenze informatiche, il fatto che abbiamo ancora troppo troppo pochi studenti che si specializzano su questa materia, il fatto che le aziende sono così parcellizzate e piccole che spesso non possono nemmeno affrontare le spese relative al rafforzamento della struttura informatica e della cybersicurezza, comportano un problema. Anche da questa direttiva e da questa attività di implementazione passano allora il rafforzamento e la qualificazione del nostro sistema imprenditoriale, della pubblica amministrazione e industriale. Ci sono poi due questioni relative al riferimento che facevo prima circa il fatto che spesso si utilizza la cornice europea per raccontare un mondo che non si riscontra nella discussione europea. prima è stata affrontata dalla collega Fregolent e dal collega Borghi in modo esemplare e riguarda la discussione sul tema del salario minimo. Noi siamo una forza politica che non ha alcun timore a dire come la pensa, anche in termini molto differenti, rispetto ai *cliché* che si utilizzano in questo Paese. Il *cliché* più attuale riguarda il fatto che, se noi attuassimo il salario minimo, avremmo tolto dalla povertà tutti i lavoratori. È lo stesso *cliché* di chi diceva che, se avessimo fatto il superbonus, avremmo risolto il problema ambientale di qualificazione delle nostre abitazioni, È lo stesso *cliché* di chi diceva che, se avessimo attuato il reddito di cittadinanza, avremmo eliminato dal balcone la povertà. *(Applausi)*. Sono paradigmi ideologici che non corrispondono alla verità. corrispondono alla verità. Hanno fatto benissimo il collega Borghi e la collega Fregolent a ricordare anche le contraddizioni che stanno in capo alla sinistra. Noi abbiamo conosciuto un sindacato che che ha ritenuto che la centralità del principio di contrattazione collettiva fosse sacrosanta. Io ho parlato tante volte, ad esempio con la collega Furlan, di questo. Oggi non è in Aula, ma sono convinta che le sue tesi fossero giuste. Ora questa discussione è invece schiacciata su un paradigma ideologico. Siamo tutti d'accordo che i salari in questo Paese siano troppo bassi. *(Applausi)*. Siamo tutti d'accordo circa il fatto che debba essere intrapresa un'iniziativa. Ma questo non può che passare passare attraverso la crescita economica ed è lì che inchiodo il Governo. È lì che chiedo a Giorgia Meloni di fare qualcosa. *(Applausi)*. Quando leggo che il ministro "Urss" per gli amici ieri si è accorto che bisogna svoltare su Ilva, rimango stupefatta. Quel collega, quel ministro, per un anno ci ha raccontato che non c'erano problemi. In ballo ci sono migliaia di posti di lavoro. Allora sì a salari migliori, no a paradigmi ideologici che, in qualche modo, limitano la nostra azione, e limitano e limitano anche un racconto vero di quello che deve avvenire in questo Paese in tema di crescita economica. Ho lasciato per ultimo il tema che tema che mi sta più a cuore. Considero questa una legislatura costituente sul tema della giustizia. Costituente significa costruire una maggioranza trasversale parlamentare

Di cosa stiamo parlando? Ci tengo a dirlo raccontando anche un fatto personale. Io ho avuto due processi, in primo e in secondo grado. Il secondo grado si è collocato quando la norma è stata cambiata.

Il racconto era stato fatto nella pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare dal punto di vista dell'accusa. È così che avviene, perché quella è una ricostruzione fattuale unilaterale dell'accusa. *(Applausi)*. È inutile che il collega Scarpinato provi tecnicamente a dare una motivazione che stia in piedi. È una ricostruzione unilaterale dell'accusa, dove non è presente

perché ho un grandissimo rispetto e una grandissima fiducia nel lavoro libero della stampa in questo Paese. E sono convinta che chiedere alla stampa di lavorare non con il copia e incolla, ma alla ricostruzione della verità, tenendo conto anche dei principi della difesa, sia un elemento di di fiducia nei loro confronti e di qualificazione del dibattito che riguarda tutti noi. È una lettura sulla quale vi prego di interrogarvi. Noi non stiamo chiedendo alla stampa di non pubblicare le notizie: noi stiamo chiedendo alla stampa di pubblicare un racconto che tenga conto del principio

la tesi più importante che dimostra che non esiste un diritto tirannico sugli altri: esiste il diritto a conoscere, ma esiste anche il diritto a tutelare le vite umane e il principio di verità.

e delle lavoratrici dai rischi derivanti da esposizione all'amianto. Ora, in conformità col piano europeo, nella lotta al cancro si doveva

cosa va fatta entro dieci anni, chiediamo di farla entro venti, cercando di mettere non il freno o

allora facciamo il mercato e la libera concorrenza dei giusti canoni e magari affrontiamo il problema della concorrenza cercando di tutelare le aziende familiari e le aziende del nostro territorio. Questa è una politica, altrimenti continuiamo ad andare in inflazione e veniamo richiamati per questo. Perché

davanti a tutti gli altri. Poi il mondo cambia, ovviamente il capitale si trasforma, i rapporti di forza cambiano e non c'è niente di male se uno cambia opinione, perché oggi la legge che fissa un minimo senza intaccare la contrattazione è un aiuto, non una gabbia.

contrattuale, il salario minimo funziona. È anche un meccanismo di recupero salariale, perché, nel momento in cui il salario minimo di fronte all'inflazione viene aumentato, anche il rapporto contrattuale è aumentato. Questo vale in in Spagna come in Germania, Paesi con cui abbiamo una certa relazione; non in Birmania, ma in Spagna e in Germania. Vale in tutti i Paesi d'Europa: è un fatto ideologico che negli altri Paesi d'Europa abbiano un minimo salariale?

e quindi si tutelano i lavoratori e le lavoratrici più deboli. È ideologica questa cosa? Per favore, si può dire che non si è d'accordo, è legittimo,

stiamo parlando della proposta di 9 euro l'ora lordi e 9 euro lordi sono pochi. Ma se pensate che ci sono quelli che ne prendono 5, chi risolve questo problema?

vale per questo, ma vale anche per le cooperative sociali e per tutte le strutture che vanno in questa direzione. È ideologica questa cosa o è un fatto concreto che risponde a un'esigenza dei lavoratori e delle lavoratrici? Per questo

intaccare il manovratore, che in sostanza è sempre il capitale. Quindi - come ho spiegato prima - per fare questa cosa bisogna spostare le risorse dal capitale al lavoro. Per fare questo bisogna spostare un po' di soldi - come si usa dire da una parte all'altra e questo significa ridurre il salario, seppur di minimo.

In questa dichiarazione di voto illustrerò per primi e con grande sintesi i principali argomenti su cui questo provvedimento interviene. Ma mi soffermerò molto più a lungo sul tema che, a torto a o ragione, ha scatenato le maggiori polemiche e l'interesse mediatico, ossia il divieto di pubblicazione integrale delle ordinanze di custodia cautelare. Il disegno di legge in esame prevede il recepimento e l'attuazione nel nostro ordinamento di ben venti direttive, di una decisione e l'adeguamento della normativa nazionale a ulteriori nove regolamenti europei. Mentre il percorso di recepimento è coerente, i contenuti sono per natura stessa delle cose non omogenei, ma tutti motivati dalla necessità di essere recepiti dalla nostra normativa. Si inizia con la direttiva sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea. Lo scopo è di aumentare il livello di cyber-resilienza e di migliorare la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Si ritiene, cioè, necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che gestiscono queste infrastrutture e che forniscono i relativi servizi essenziali. Vengono quindi adeguate alla normativa italiana le norme sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Viene prevista l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali. Inoltre, viene recepita la direttiva sugli acquirenti e gestori di crediti deteriorati. Viene recepita anche la direttiva sulla protezione dei lavori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Entra nel nostro ordinamento anche l'idea di rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Sono previste nuove norme per commercializzare le apparecchiature radio installate sugli aeromobili. Viene modificata la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità che attribuisce a Consob il compito di coordinare le disposizioni nazionali. È apprezzabile anche la direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate. Vengono stabilite a disposizioni anche sulla collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione dell'Unione europea. Detto ciò in ordine agli interventi di carattere generale - come le avevo anticipato, signor Presidente - mi soffermerò per il residuo tempo a mia disposizione sul divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare. Con questa modifica introdotta alla Camera, che noi confermiamo, si è sostanzialmente ripristinato il divieto che era vigente ante 2017; divieto che peraltro fino a quel momento non aveva mai creato problemi né scatenato nessuna indignazione o dubbi di costituzionalità. Quindi, non comprendo e non giustifico il caso mediatico che si è voluto a tutti i costi creare in queste settimane. Il tutto - mi pare - si basa su un grande equivoco. Il divieto approvato in prima lettura alla Camera è semplicemente una norma di buon senso e di civiltà giuridica, che ha il solo scopo di evitare che in futuro sui giornali finiscano come purtroppo è accaduto in passato tante volte - le intercettazioni integrali riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, danneggiando spesso irrimediabilmente l'immagine o la reputazione di chi in quelle intercettazioni è coinvolto o è citato. Quello della pubblicazione dei virgolettati delle intercettazioni è un fenomeno deprecabile che non accade in alcun altro Paese al mondo, tranne l'Italia. Proprio a questa vistosa eccezione si è voluto porre rimedio con la norma in esame. Spesso i virgolettati contengono battute ironiche, doppi sensi, espressioni gergali talora anche di cattivo gusto o addirittura scurrili, che però, decontestualizzati, sono finalizzati solo alla pubblica denigrazione dei soggetti coinvolti, più che alla prova di una qualche responsabilità penale. Gli esempi di linguaggio colorito riportati in passato testualmente sui giornali al solo scopo di esporre alla gogna mediatica i soggetti coinvolti sono innumerevoli. Ieri ne ho citati un paio, i primi che mi sono venuti in mente, ossia quello della «sguattera del Guatemala» e quello riferito alle battute, molto più recenti temporalmente, del presidente Zaia soggetto non indagato - sul collega senatore Crisanti - parimenti soggetto non indagato - nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità veneta. Ieri, replicando alla mia dichiarazione di voto, il senatore Scarpinato, che adesso non vedo in Aula - magari ci penserà lei, signora Presidente, a riferire le mie argomentazioni, le mie controdeduzioni - ha parlato di inconsistenza giuridica degli esempi da me citati, sostenendo che non erano pertinenti, perché a suo dire si riferivano alla disciplina ante riforma Orlando, che a suo giudizio invece avrebbe ovviato a quegli eccessi. il senatore Scarpinato ha errato: se l'argomento poteva essere fondato relativamente all'inchiesta Tempa Rossa della procura di Potenza risalente al 2016, non lo era certamente per la recentissima inchiesta della sanità veneta, che invece è dell'anno scorso, quando da tempo era vigente la riforma Orlando e a cui ha dato ampio risalto, per esempio, la trasmissione televisiva «Report». Cosa rimane di queste inchieste a distanza di molti anni o di qualche tempo? Dal punto di vista giudiziario direi molto poco;

Per questo mi paiono incomprensibili le ragioni dello *strepitus* mediatico che si è acceso su questa norma, che peraltro non vieta affatto ai giornalisti di fare il loro lavoro, né impedisce loro di dare notizie.

per farci capire da chi ci sta ascoltando da casa - potremmo definire il cosiddetto copia e incolla totale o parziale del provvedimento. Pertanto, in futuro al giornalista non verrà vietato di parlare dell'ordinanza di custodia o dei suoi contenuti, di illustrarla anche nei dettagli, di commentarla, ma dovrà farlo mediante una sintesi, una parafrasi, un riassunto più o meno critico. In questo modo, tra l'altro, si potranno valutare le sue qualità professionali, le sue capacità argomentative di ragionamento e anche il rispetto delle norme deontologiche. Era troppo semplicistico limitarsi al copia incolla. In futuro i bravi giornalisti non avranno alcun problema a continuare a svolgere il loro lavoro e a continuare ad assicurare la completa informazione dei lettori; probabilmente, invece, troveranno una difficoltà i cosiddetti velinari delle procure, quei giornalisti di cronaca che magari non posseggono una penna facile o una scrittura fluente, ma piuttosto sono adusi alle relazioni privilegiate con avvocati, uffici di polizia giudiziaria, di procura, insomma alle

Nel Regno Unito, in Lussemburgo, in Svizzera, in Germania vigono norme a tutela degli indagati in materia di pubblicazione degli atti giudiziari ben più stringenti di quelle oggi all'esame dell'Assemblea e che andiamo ad approvare. mi consenta un'ultima annotazione. Negli ultimi giorni era stato dato ampio risalto sulla stampa alla richiesta del MoVimento 5 Stelle di votare a scrutinio segreto l'articolo 4 del testo in esame che conteneva, appunto, la presunta legge bavaglio. Poi, alla chetichella, questa richiesta è stata ritirata, come è stato fatto ieri per quanto riguarda il voto finale del cosiddetto disegno di legge Nordio sulla riforma della giustizia. Evidentemente l'esperienza della settimana scorsa è servita a far capire che sui voti segreti questa maggioranza aveva più voti che nei voti palesi. Signora Presidente, a buon intenditor poche parole.

siamo alle battute finali di un percorso più o meno lungo e travagliato. Parliamo di temi importantissimi per la Nazione, perché - come tutti ben sappiamo le normative e le politiche dell'Unione europea ormai entrano appieno in tutta la normativa nazionale. dare massima importanza e rilevanza a una delle due leggi che, ai sensi della legge n. 234 del 2012, ci permette di aprire e di dialogare con l'Unione europea, e spesso - mi dispiace sottolinearlo, signor Presidente, magari lanciamo un messaggio al Ministro e a chi governa questi processi - bisognerebbe dare maggior rilievo e importanza a questi momenti. Mi dispiace intervenire in un'Aula praticamente vuota, questo dà anche la cifra dell'interesse e della sensibilità di un ramo del Parlamento a importantissime tematiche.

denota e dà la cifra precisa della prontezza di quelli che si dichiaravano in campagna elettorale, nel settembre 2022, pronti a governare e dopo un anno e mezzo ci portano delle norme palesemente scadute. *(Applausi)*. Complimenti: state dimostrando agli italiani che vi vedono e vi seguono che siete in ritardo su tutta la linea e i dati e i documenti lo dicono a chiare lettere. Pertanto, per il suo tramite, Presidente, mi rivolgo ai membri del Governo e al ministro Fitto: abbiamo trattato, in questa legge di delegazione, vari argomenti, alcuni portati al suo interno con delle forzature procedurali. Già ieri in dichiarazione di voto ho messo in evidenza quello che si è consumato nell'altro nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera dei deputati, con l'attuale articolo 4. Ribadisco che quella è una forzatura procedurale che andava bloccata in quella sede; invece qui al Senato ce la siamo ritrovati senza poter neanche chiedere l'inammissibilità, perché andava fatto in quella Camera. È stato inserito in una legge di delegazione europea un argomento citando e richiamando una direttiva che era già stata attuata con un decreto legislativo. Già nel 2021 la Commissione europea non ha messo in rilievo niente e, pertanto, non c'erano neanche i presupposti procedimentali per portare in Aula un tema così importante. Chiamatela come volete, legge bavaglio? Lascio a chi ha fatto dei commenti puntuali, ai colleghi che sono più esperti di me in materia, che hanno argomentato ampiamente su questo tema.

L'Italia e il Governo si vantano - ma la Meloni in particolare si vanta - dicendo che, quando va lei in Europa, si aprono le porte ed i portoni. E questi sono i risultati? Con il patto di migrazione ci hanno di nuovo preso a sberle. Il patto di migrazione non andrà a modificare il Trattato di Dublino, e venga detto in maniera chiara. Cosa ci ha portato, dunque, questo patto, grazie al grande lavoro di mediazione di questo Governo? Il nulla. In buona sostanza, noi eravamo e rimaniamo Paese di primo approdo, che è il principale problema legato al Trattato di Dublino. In più, vi è l'aggravante che ora avremo l'onere di

Torniamo a quelli che sono i flussi secondari. Non abbiamo risolto niente. Anzi, ora Stati come Francia e Germania potranno rinviare in Italia i migranti con una mera comunicazione, quando prima dovevano provvedere ad una notifica. Ora basta una mera comunicazione e rimanderanno indietro anche

Nel pomeriggio tratteremo anche la questione Albania: deportando 3.000 disperati in Albania, risolveranno i problemi. Pertanto, il pacco sulla migrazione è bello che consumato. Nella migliore delle ipotesi, con i flussi secondari, se, nel caso di redistribuzione, gli Stati non vorranno, potremo chiedere un indennizzo, dal momento che non c'è alcun sistema obbligatorio di redistribuzione. Bravi! Complimenti! Andiamo all'altro pacco, al pacco di stabilità. Anche qui, toni trionfalistici fino a qualche settimana fa, ma ora anche questo pacco si è consumato. I sovranisti *de noantri* - come dicono a Roma - hanno prodotto cosa? Super rigorismo. Siamo rimasti sul super rigorismo, senza riuscire a scardinare nulla di quelli che erano i veri problemi legati al Patto di stabilità. Pertanto, il rigido parametro del 3 per cento del *deficit* in rapporto al PIL è rimasto per cento del debito in rapporto al PIL. Signori, quali sono le conquiste che avete ottenuto in Europa? Ditecelo, perché, ogni volta che si chiude un procedimento, poi i fatti vi smentiscono. Noi, quelli meno bravi, con il Governo Conte siamo riusciti a ottenere 209 miliardi con il PNRR. Voi cosa avete ottenuto? Noi siamo riusciti a cambiare qualcosa che sembrava inimmaginabile poter cambiare. Parlo di debito comune europeo. Col Next generation EU, noi siamo riusciti a portare una novità.

un indirizzo chiaro a quelle che sono le criticità di quel processo, nel quale mancano dei sistemi di valutazione puntuale delle emissioni e, di conseguenza, per andare a valutare anche emissioni di comparti come quello dell'edilizia. dell'edilizia. Passo al tema legato al salario minimo. Come è stato ampiamente detto, quella tematica importantissima è stata derubricata dal Governo mettendola al punto quattro dell'allegato A.

mettendo in chiaro quali erano gli obiettivi. Non ritorno sul tema, che è stato ampiamente trattato; non c'è alcuna incompatibilità tra il salario minimo e la contrattazione collettiva nazionale, che palesemente ha fallito in questa Nazione. Diamoci una mano per risolvere i problemi del lavoro povero, perché questo Governo ha dimostrato di essere bravo e vicino ai grandi gruppi industriali e invece molto distratto e contrario di fronte a chi non riesce ad arrivare alla terza settimana, tante parti di questo disegno di legge di delegazione. Presidente, mi avvio alla conclusione e dichiaro così il voto di astensione, con grande rammarico. La legge di delegazione europea deve o dovrebbe essere uno strumento utile ad evitare che la Nazione continui a pagare centinaia di milioni, perché questo è quello che ci costa ogni anno, oltre 100 milioni di euro l'anno. Finora, al 2022, stiamo parlando di quasi un miliardo di euro dato per le sanzioni dell'Unione europea. Pertanto confermo e ribadisco il voto di astensione. Si spera - e inviamo tale messaggio al ministro Fitto - di portare per tempo questa importantissima legge di delegazione europea e di evitare i decreti, come ha fatto per la legge europea. Presidente, gentili colleghe senatrici e colleghi senatori, vorrei *in primis* ringraziare i colleghi qui seduti, perché questa è una dimostrazione di maggioranza che convintamente vuole approvare questo disegno di legge di delegazione europea. Siamo finalmente alla fine di questo lungo e importante *iter* e sembra che siamo in ritardo, perché stiamo per approvare la relazione consuntiva 2022 e quella programmatica 2023. Ma nella proposta di risoluzione di maggioranza che è stata presentata chiediamo al Governo di avere al più al più presto la relazione consuntiva 2023, la relazione programmatica 2024 e la legge di delegazione europea, in cui abbiamo chiesto di inserire direttamente le problematiche relative alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo *ex* articolo 260, che già danno luogo al pagamento di sanzione pecuniarie, e alle procedure di infrazione che mano a mano comportano meno problematiche economiche. Questo è sicuramente un segnale di attenzione e sappiamo che il ministro Fitto ci sta lavorando. Tuttavia faccio presente che in questo provvedimento andiamo a recepire sette regolamenti e sedici direttive, ma non andiamo a sanare infrazioni, perché lo abbiamo già fatto con il decreto-legge infrazioni a luglio 2023. questo disegno di legge di delegazione europea andiamo a prevenire costi per lo Stato e andiamo a prevenire le infrazioni. Fra gli emendamenti che sono stati accolti, anche alla Camera, ci sono emendamenti sulla giustizia e sulla parità salariale e c'è un ordine nel giorno sulla cybersicurezza. Questo è un tema molto importante, che affrontiamo nell'articolo nell'articolo 3, dove andiamo a recepire la direttiva 2022 sulla cybersicurezza, che è uno dei temi importanti del PNRR per garantire la sicurezza dei dati delle persone, specialmente dei nostri giovani, che usano costantemente i *social* e il mondo Internet. Si tratta di un tema importantissimo; la scorsa settimana abbiamo ricordato il Safer

il Governo a valutare l'opportunità di togliere la discriminazione che ancora c'è nel mondo della scuola per il personale docente di ruolo e quello messo a ruolo, così pure come i *benefit* per il buono docenti, anche per i supplenti. Sicuramente è importante anche quello che viene inserito nell'articolo 11, relativo alla rendicontazione ambientale per una transizione verde che sia consapevole e socialmente sostenibile. Quindi no all'agenda Timmermans e no all'agenda Greta, come penso abbiano dimostrato le proteste degli agricoltori, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Serve un'applicazione della transizione verde a livello nazionale, che tenga conto del diritto dei lavoratori, delle imprese, del nostro sistema economico e dell'autonomia strategica. Tutelare l'agricoltura italiana e la dieta mediterranea vuol dire tutelare la nostra cultura, difendere le nostre tradizioni e le nostre produzioni; tutelare gli agricoltori vuol dire tutelare noi stessi da incendi, da alluvioni e dalla crisi alimentare. È sicuramente importante. Un segnale è stato dato anche con l'accoglimento dell'ordine del giorno per introdurre il calcolo della *carbon footprint*, della *water* *footprint* e dell'*ecological footprint*, anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA. L'articolo 16 riguarda il recepimento del regolamento europeo concernente i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi derivati da cripto-attività relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il finanziamento del terrorismo. Questo sicuramente è un altro importantissimo atto per il livello di sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini. Abbiamo espresso invece un parere contrario alla proposta emendativa sul salario minimo e vorrei spiegare perché, addentrandomi direttamente in questa problematica che già avevamo affrontato anche nella discussione generale. La direttiva europea 2041 del 19 ottobre ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per tutti i lavoratori in Europa: 21 dei 27 Paesi europei hanno un salario minimo garantito, ma sei - l'Italia, l'Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia - determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva delle retribuzioni. Dall'entrata in vigore della direttiva, abbiamo due anni per poterla recepire. Perché dunque è strumentale il richiamo alla direttiva europea e dire che ce lo chiede l'Europa? Perché proprio la direttiva europea non ha previsto, come si vorrebbe far credere, un obbligo di introduzione del salario minimo nei Paesi che ancora non lo prevedono, ma impone agli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva è insufficiente, di prevedere un quadro per la contrattazione collettiva e di istituire un piano d'azione per promuoverla, per garantire che i salari minimi siano fissati ad un livello adeguato. L'Italia è fra i Paesi europei con la più alta copertura contrattuale, già oggi superiore a quanto la direttiva in discussione indica come obiettivo per il futuro. Quindi non c'è alcuna procedura di infrazione e non ce lo chiede l'Europa. Esiste una proposta di legge dei 5 Stelle, già discussa alla Camera, su cui il Governo si è espresso con un emendamento interamente sostitutivo a firma del Capogruppo della Commissione lavoro; si intende delegare il Governo a garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva ed emanando, entro sei mesi dalla data in vigore della legge, dei decreti attuativi per assicurare ai lavoratori trattamenti giusti, per contrastare il lavoro sottopagato e stimolare il rinnovo dei contratti collettivi. C'è un altro emendamento che è stato bocciato che è quello relativo alla direttiva Bolkestein, la famosa legge sui balneari. È stato bocciato, perché esiste già una procedura di infrazione - è vero - però esiste un tavolo nazionale ed esiste anche una contrattazione con l'Europa, per cui non possiamo minimizzare con l'approvazione di un emendamento e scavalcare la contrattazione che il Governo sta portando avanti con l'Europa. Quindi, come avrete capito, c'è direttamente un disegno all'interno di questa legge di delegazione europea per prevenire queste procedure di infrazione. Il dibattito vero verte appunto sul ruolo dell'Unione europea e sul suo impatto sulla vita dei cittadini e delle imprese. Purtroppo in questi anni, specialmente con l'ultimo Parlamento europeo, sono state più le imposizioni che i miglioramenti a tutela degli Stati europei, dei cittadini, delle imprese europee, specialmente piccole e medie imprese (come quelle che compongono il nostro tessuto imprenditoriale), dell'agricoltura e della nostra concorrenzialità. Ecco, tutto il mondo produttivo si è accorto, e così pure i cittadini, che serve un cambiamento in Europa e sicuramente il vento del cambiamento sta arrivando e lo vedremo a giugno. Non si può continuare con il *mood* «ce lo chiede l'Europa». L'Europa deve tutelare di più i propri cittadini, valorizzare le diverse culture, differenze e produzioni e non deve essere usata come uno strumento con il quale solo alcuni Stati riescono a potenziare la loro egemonia.

alla responsabilità che abbiamo come partito e come Paese nei confronti delle istituzioni europee. Sappiamo che l'Italia è tra i Paesi più in difficoltà per esempio sul fronte delle procedure di infrazione. Ad interrogarvi sulla condotta seguita dovreste essere voi, colleghi della maggioranza, con un disegno di legge di delegazione europea in grave ritardo. andava presentata entro il 28 febbraio, ma del 2023, un anno fa. Un ritardo che si inserisce nel contesto del *deficit* politico sostanziale di questo provvedimento, che è usata dal Governo per difendere le sue norme di parte e non condivise. Noi che sempre abbiamo condiviso la necessità del provvedimento, intendendolo di interesse nazionale, denunciamo e ci opponiamo a un simile snaturamento della legge che dovrebbe servire a inserire nel nostro ordinamento norme attuative delle nuove direttive UE. La lesione che viene inferta ai cittadini nel loro diritto all'informazione rappresenta da sola un tale *vulnus* da imporci un'opposizione fermissima. La legge bavaglio non è però il solo punto critico di un provvedimento che presenta troppe zone d'ombra e troppe ambiguità, come è il caso del recepimento della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea, volta a migliorare le condizioni di lavoro e di vita all'interno dell'UE, riducendo le disuguaglianze retributive attraverso la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, l'adeguatezza dei salari minimi legali e l'accesso effettivo delle lavoratrici e dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo. Solo qualche settimana fa avete affossato la proposta di legge sul salario minimo, presentata da quasi tutte le opposizioni, che viene richiesta trasversalmente da centinaia di migliaia di cittadini che hanno apposto la loro firma su questa richiesta. Cittadini che non vivono certo la realtà di questi palazzi, ma quella reale, che si pongono il problema di come riempire il carrello della spesa, come arrivare a fine mese, come affrontare il pagamento delle bollette, l'affitto o la rata del mutuo, come dare ai propri figli la possibilità sacrosanta di poter studiare poter studiare e così via. Siccome non avete voluto decidere, l'avete sostituita con una delega in bianco al Governo, senza alcuna effettiva possibilità di confronto. Un atteggiamento davvero riprovevole. Il salario minimo per noi del Partito Democratico è un traguardo non rinunciabile e lo è per qualsiasi Paese voglia definirsi civile. *(Applausi)*. Altro aspetto significativo di questo provvedimento è la direttiva riguardante il rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro e per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e le garanzie di accesso a strumenti di tutela. Altrettante significative sono la direttiva volta al miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate o ancora la direttiva che interviene in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori e delle lavoratrici contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Particolare importanza ha anche il recepimento delle direttive in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Sono tutti temi sui quali purtroppo è ormai tristemente nota la posizione di questa maggioranza e di questo Governo. Ci sono norme volte a tutelare i nostri cittadini e le pubbliche amministrazioni rispetto ai rischi derivanti dagli attacchi *cyber* e *online*, volte a rafforzare la cybersicurezza nel nostro Paese. Anche in tal caso, senza fare propaganda, dico che abbiamo visto quanto sia semplice, facile o possibile bucare la rete telefonica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. quanto sia essenziale rafforzare la tutela delle pubbliche amministrazioni e dei nostri cittadini rispetto all'utilizzo dei dati sensibili che circolano nel nostro Paese. I colleghi Verini e Sensi hanno parlato ampiamente dell'emendamento Costa, che vieta di fatto ai giornalisti la pubblicazione, anche per estratto, delle ordinanze di custodia cautelare. Ciò non corrisponde alla direttiva europea 2016/343, che stabilisce la necessità di di rispettare il principio di presunzione di innocenza (diritto peraltro sacrosanto), ma che non si occupa di limitare la pubblicazione di atti di indagine. Al contrario, sottolinea la necessità di salvaguardare la libertà di stampa ed è inoltre in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sono concetti, questi, espressi dal presidente dell'ordine dei giornalisti durante le audizioni alla Commissione del Senato. La pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare che non sono segrete fa parte di quella libertà di informazione che determina per i cittadini il diritto di conoscere l'attività della magistratura, attività peraltro ancora autonoma, e speriamo tale rimanga. La democrazia, signora Presidente, ha regole molto precise, ma non passa certo attraverso l'autarchia governativa. Quest'ultima riporta ad altri tempi, di cui è inutile ricordare gli orrori e i fallimenti. In effetti, ci porta anche verso altri Paesi, che l'autonomia che l'autonomia della magistratura l'hanno abolita e che calpestano il diritto; Paesi come l'Ungheria di Orbán, che possono permettersi di fare la voce grossa col Governo italiano perché sanno di non avere conseguenze, anche se incarcerano e umiliano pubblicamente una nostra concittadina. Allora, ci sono italiani che valgono di meno? *(Applausi)*. Signora Presidente, noi continuiamo a chiedere a questo Governo di non sottrarsi al confronto su temi di così cruciale importanza, come il nostro rapporto con l'Unione europea e il ruolo che che vogliamo avere in Europa. Ma non ci stupiamo più di nulla, nemmeno del ritardo col quale questa maggioranza e questo Governo stanno agendo in questo momento su un altro provvedimento, ed è bene ribadirlo anche in questa sede. C'è uno strumento che solo l'Italia, tra i 27 Paesi, non ha recepito, né ha approvato

Cogliamo ancora una volta l'occasione per dire che la riforma di uno strumento che esiste dal 2012 migliorerà semplicemente le tutele dei risparmiatori italiani ed europei. C'è infatti una norma, il cosiddetto *backstop*, che consente di sostenere con risorse del MES il Fondo unico per le risoluzioni bancarie, ossia per le crisi bancarie, consentendo al MES di intervenire in caso di crisi di istituti bancari, tutelando i risparmiatori e i consumatori italiani ed europei. Voi state bloccando questa norma ancora una volta, decidendo di non decidere, rispetto alla ratifica della modifica al trattato sul MES. *(Applausi)*. Siamo l'unico Stato a non averlo ancora fatto, in un contesto nel quale, peraltro, l'Italia rischia di perdere credibilità sui tavoli europei di Bruxelles. Questo di oggi è un provvedimento importante. Recepire direttive fondamentali, come quelle ricordate, vuol dire contribuire a migliorare il processo di integrazione europea e a migliorare le tutele e le garanzie dei nostri cittadini, che il livello europeo è quello più adeguato ed è l'unico in grado di consentirci di affrontare le sfide e le criticità del nostro tempo. Gli Stati nazionali da soli non sono in grado di rispondere alle criticità del nostro tempo, di dare risposte ai nostri cittadini. Questo è il punto centrale, centrale, politico, su cui poniamo l'attenzione. Invitiamo davvero tutte le forze politiche italiane - l'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea - a non fare passi indietro. L'Europa è la nostra casa comune. L'Europa è l'unico livello istituzionale e politico in grado di difendere davvero le nostre comunità e i nostri cittadini nei prossimi anni, di fronte alle sfide drammatiche che abbiamo dinanzi nel nostro tempo. Lo vediamo: sono sfide geopolitiche, sfide legate ai conflitti, sfide legate alla pandemia, sfide legate all'energia, legate al rafforzamento delle tutele sociali. Per tutto questo, e concludo, abbiamo bisogno di un'Europa più forte, di un'Europa rinnovata, di un'Europa davvero politica ed è questo il lavoro che dovremmo fare. Guai ad andare indietro, guai a ritornare indietro guai a ritornare indietro alle piccole e vecchie patrie, perché danneggeremmo in modo irreparabile il futuro dei nostri cittadini.

per il ruolo che ha svolto in Commissione, riconosciuto anche dalle opposizioni, avendo saputo ascoltare e ricomprendendo anche molte delle osservazioni che venivano dalla minoranza, portando il testo in Aula così com'è, insieme alla collega Murelli, relatrice delle relazioni di accompagnamento. Voglio anche ringraziare il sottosegretario Siracusano, sempre molto presente in Commissione,

maggioranza e minoranza e per aver saputo offrire la disponibilità del Governo ad intervenire su ognuna di queste fattispecie. Noi oggi approviamo una legge che, come sappiamo tutti, permette il

e siamo più o meno tutti sulla stessa linea. È inutile nasconderci dietro un dito e sottolineare quello su cui non siamo stati d'accordo e su cui abbiamo anche visto in quest'Aula un'evidente distinzione. La prima è quella che viene definita legge bavaglio. Come abbiamo già detto, se esiste questa legge bavaglio, allora dobbiamo dire che fino al 2017 la stampa italiana è stata imbavagliata, perché questa norma è stata introdotta nel 2017. La stampa italiana ha avuto il sentore di non potersi esprimersi liberamente? Non mi pare. Allora ogni tanto bisogna avere il senso della realtà oserei dire - anche il senso del ridicolo quando affermiamo certe cose e avere, visto il tema, un senso di giustizia. C'è chi l'ha detto prima di me: noi stiamo parlando di un'ordinanza cautelare, che è un'ordinanza di parte. È l'ordinanza emessa da chi giustamente fa il proprio lavoro come magistrato inquirente, ma non ma non c'è la parte della difesa. Permettetemi di dirlo, se abbiamo ancora a cura il garantismo e la voglia di stare dalla parte di chi viene accusato fino a prova contraria. perché accadono delle cose in questo Paese molto più gravi, anche quando andiamo oltre questo livello e questo grado. Lo voglio dire anche per ricordare una situazione anche anche ha visto coinvolto il nostro capogruppo al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, che due anni fa è stato infangato in ogni luogo sui giornali e sulle televisioni per una presunta - per noi sempre, perché siamo garantisti - *lobby* nera. Qualche giorno fa il primo grado della magistratura ha detto: di che cosa parliamo? Non c'è nulla. Dove stanno i giornalisti liberi e indipendenti, che hanno ridato a Carlo Fidanza la sua dignità? Dove stanno i giornali e le televisioni che hanno potuto sottolineare questo aspetto? Se questo non avviene su casi così importanti e così gravi, figuriamoci su un'ordinanza cautelare. Allora di questo noi oggi parliamo, perché se noi riconosciamo a tutti i giornalisti il diritto di indagare e di scrivere, dobbiamo anche ricordare che che hanno un dovere, quello di pensare, scrivere e anche evitare che alcune persone finiscano in un tritacarne, da cui poi - guarda caso - non sanno più come uscirne, non tanto per motivi legali, ma per motivi di informazione. Veniamo a un altro aspetto, quello che abbiamo ricordato come il salario minimo. Nel provvedimento, quando si parla di salario minimo e quando quindi l'Unione europea ci dice di essere attenti a questo aspetto, non si dice che la proposta del salario minimo deve essere quella che ha in testa il Partito Democratico o il MoVimento 5 Stelle, perché è invece un'altra cosa. cosa. Il MoVimento 5 Stelle ha avuto cinque anni per fare il salario minimo e non l'ha fatto *(Applausi)*. Il Partito Democratico ha avuto dieci anni per fare il salario minimo e non l'ha fatto. Proprio adesso, in questo momento specifico, però c'è necessità del salario minimo? Fino ad ora non ce n'era bisogno? Proprio nel momento in cui Giorgia Meloni varca la soglia di Palazzo Chigi,

Come si suol dire, non era un «impegna», ma una raccomandazione. SCURRIA ricordiamo le parole della CGIL e di alcuni sindacati sulla contrarietà al salario minimo, che oggi invece diventa battaglia di civiltà. In Europa c'è il salario minimo laddove non c'è una contrattazione collettiva così precisa e così puntuale come avviene in Italia. Si è parlato di alcuni esempi anche in Europa.

retribuzione che i contratti collettivi nazionali garantiscono. Lo so che questo è un vizio storico e culturale della sinistra, ossia quello di appiattire e di livellare sempre verso il basso le retribuzioni, ma noi abbiamo un'altra impostazione. Si citava la Germania, ma in c'è una contrattazione collettiva molto bassa; per questo c'è spazio anche per altri esperimenti. Nella sperimentazione che c'è in Germania, in alcuni contratti che prevedono un rapporto diretto tra datore di lavoro e lavoratore

punta a migliorare la condizione di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori, al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle diseguaglianze retributive. Ma la direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante i contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Questo è quello che troviamo nella direttiva europea ed è ciò che noi recepiamo attraverso il nostro intervento sul disegno di legge di delegazione europea. Concludo, signor Presidente. Fino a qualche tempo fa le leggi di delegazione europea passavano in maniera quasi anonima in quest'Aula. Adesso questa legge è diventata centrale e se n'è discusso anche grazie anche grazie al peso che questo Governo dà all'aspetto europeo e al peso che l'Italia ha in Europa. Qualcuno ha fatto qualche umorismo prima sulla nostra capacità di presenza in Europa e su quello che il Governo Meloni sta facendo in quella buona pace di tutti i nostri colleghi eravamo pronti a governare e lo stiamo dimostrando attraverso la diminuzione delle infrazioni che abbiamo raggiunto in questo Paese, attraverso l'aumento dei posti di lavoro, attraverso il recupero dell'evasione fiscale. Ma non lo diciamo noi: voglio tranquillizzarvi e rassicurarvi per quello che riguarda l'immagine italiana nel mondo, perché di successo diplomatico-migratorio di Giorgia Meloni parla «Le Monde»; dell'influenza che Meloni sa esercitare in Europa parla il «The New York Times»;

le Commissioni riunite 1a e 3a sono state autorizzate a convocarsi alle ore 14 per il seguito dell'esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Conseguentemente, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta riprenderà alle ore 16,15 con l'esame di tale disegno di legge. I tempi della discussione sono stati ripartiti per complessive quattro ore: tre ore per i Gruppi e un'ora per i tempi tecnici di votazione, escluse le dichiarazioni di voto finale. La seduta di oggi terminerà alle ore 20,30. L'esame della ratifica, se necessario, potrà proseguire domani mattina. Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario dei lavori della settimana corrente. La Conferenza ha convenuto altresì all'unanimità sulla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge sul Monteverdi Festival di Cremona. La Conferenza dei Capigruppo tornerà a convocarsi mercoledì 21 febbraio, alle ore 14. **Calendario dei

di audire urgentemente il ministro Fitto. Abbiamo chiesto già da diverse settimane che il ministro Fitto venga a relazionare in Aula sulla rimodulazione del PNRR. A distanza di un mese e mezzo dall'approvazione in Consiglio europeo, i Comuni italiani sono ancora in attesa di sapere che ne sarà degli 11 miliardi di progetti finanziati dai fondi del PNRR

che venga il prima possibile, certamente entro la settimana prossima, perché il Parlamento non può più attendere di sapere come è stato rimodulato il PNRR, come verranno spesi quei fondi, come verrà data risposta ai Comuni italiani che sono in attesa di sapere che fine hanno fatto i fondi per i progetti per 11 miliardi di euro che sono di Prego

che è accaduto negli ultimi sei mesi, che ha certamente importanza, ma segue il suo *iter* normativo *standard*, perché è obbligo del Ministro relazionare sulla semestrale. Noi chiediamo di capire qual è la situazione in atto, perché leggiamo anche dalla stampa

Signora Presidente, vorrei riferire all'Assemblea che abbiamo concluso i nostri lavori alle ore 16, come era stato deciso in Conferenza dei Capigruppo.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

Signora Presidente, questo accordo (e il disegno di legge che lo ratifica) istituisce, con il fine dichiarato di intervenire sulla cosiddetta emergenza immigrazione, un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, peraltro esterno all'Unione europea, che prefigura la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri. Il disegno di legge in esame presenta - a nostro avviso - evidentissimi profili di illegittimità costituzionale, in particolare in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione e si pone in contrasto anche con delle norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea. Per questo motivo abbiamo posto una questione pregiudiziale di costituzionalità. Come è stato efficacemente detto dal dottor Schiavone nel corso delle audizioni, si prefigura la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri, in cui avremo addirittura una sezione penitenziaria con il distaccamento di un contingente della Polizia penitenziaria italiana. E come è stato chiarito anche da un altro degli auditi, il costituzionalista Bonetti, il Protocollo italo-albanese, alla luce delle disposizioni legislative nazionali di esecuzione e delle altre norme legislative nazionali vigenti in esse richiamate, configura una cessione temporanea per cinque anni dell'uso di una porzione del territorio albanese da adibirsi all'allestimento e alla gestione di due centri, un punto di crisi *hotspot* (un CPR), e una sezione penitenziaria, i quali saranno adibiti allo svolgimento di operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3.000 stranieri l'anno soccorsi in acque internazionali che vi saranno portati da navi militari italiane, nelle quali saranno soggetti alla legislazione italiana. Il primo dato è che si prevede l'applicazione extraterritoriale di norme dell'Unione europea che però non è consentita dal diritto europeo. In Albania, Paese attualmente non facente parte dell'Unione, non può infatti trovare applicazione il diritto dell'Unione europea, come peraltro valutato preliminarmente dalla stessa Commissione. Nel testo del Protocollo non c'è menzione né dell'esclusione delle persone minori e vulnerabili dal trasferimento in Albania e nemmeno delle procedure per il corretto accertamento dell'età e la tempestiva individuazione e presa in carico delle vulnerabilità prima dell'arrivo o all'interno dei centri, fatto che si porrebbe in aperta violazione della direttiva n. 32 del 2013 dell'Unione europea. È utile ricordare che il personale delle navi non può operare valutazioni allo scopo di autorizzare sbarchi selettivi e non è inoltre chiaro se i centri da realizzarsi in Albania saranno destinati alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e, in particolare, alle procedure di frontiera o al rimpatrio, ma alle persone condotte nei centri sarebbe impedito di uscire, subendo di fatto un regime di detenzione automatica e prolungata, senza che però intervenga una qualche chiara base legale. Inoltre, non è garantito il diritto di difesa. Non si comprende cioè come si potrà determinare la competenza del giudice che dovrà convalidare il trattenimento, non si comprende come sarà possibile, per i trattenuti, presentare tempestivamente un ricorso e da questo punto di vista appare evidente la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nella pratica, cioè, come è stato evidenziato anche da importanti organizzazioni come Amnesty International, secondo il diritto internazionale il godimento della libertà personale deve rimanere sempre e comunque la condizione di base di ogni individuo. Qualsiasi restrizione al diritto alla libertà deve essere eccezionale e deve basarsi su una valutazione caso per caso della situazione personale di ciascuna persona migrante e richiedente asilo interessata. La valutazione individuale deve essere relativa alla salute fisica e mentale delle persone migranti irregolari o richiedenti asilo, nonché a fattori come la loro storia personale, l'età, le condizioni di salute, la situazione familiare, eventuali esigenze specifiche. Politiche, invece, di detenzione generalizzate o automatiche sono, dal nostro punto di vista, del tutto arbitrarie perché non si basano su una valutazione individualizzata della necessità e della proporzionalità della misura di detenzione, che sono evidentemente capisaldi della nostra cultura giuridica. Le persone rifugiate richiedenti asilo, i migranti devono già affrontare ostacoli per fare ricorso contro il il rigetto delle domande di asilo e le decisioni di detenzione, soprattutto quando sono confinate negli *hotspot* oppure detenute nei centri di rimpatrio in Italia. E si tratta molto spesso di ostacoli di natura finanziaria, di natura linguistica o di natura burocratica. È quindi inaccettabile che queste barriere vere e proprie diventino sempre più insormontabili per le persone detenute dalle autorità italiane in Albania. Inoltre, il dato secondo il quale l'accordo tra Italia e Albania non prevede la possibilità per le persone di essere rilasciate dai centri, se non attraverso il trasferimento in Italia, pone esso stesso il rischio che le persone che vincono i ricorsi contro il trattenimento debbano, di fatto, rimanere in detenzione nelle more dell'organizzazione del loro trasferimento, che potrebbe, evidentemente, richiedere un periodo di tempo assolutamente significativo.

Signor Presidente, noi poniamo una questione di legittimità costituzionale, perché siamo convinti che la legge debba garantire uguali diritti, uguali doveri, uguali garanzie per tutti i cittadini, indipendentemente dal colore della loro pelle, dalla razza e dalla provenienza. Pensiamo che questo sia il fondamento del diritto. Pensiamo che questo sia quello che ha reso la nostra civiltà una civiltà avanzata, una civiltà che ha

Tante persone si stanno chiedendo il motivo di questo provvedimento. Qual è la necessità che ha spinto il Governo a procedere con un provvedimento di questo tipo? Ogni legge

da una visione della convivenza civile. Ogni legge, poi, ha anche una funzione pedagogica. Fin dagli antichi tempi, sant'Isidoro di Siviglia nel Settimo secolo e san Tommaso d'Aquino parlavano del fatto che le leggi inducevano gli uomini alla virtù, che hanno proprio questo scopo, di indurre gli uomini alla virtù, al bene, ai comportamenti corretti, ai comportamenti che edificano la società. è una legge non pedagogica. È una legge pericolosa, che porta l'uomo al vizio. Ora, io mi domando e domando a tutti noi, se vogliamo essere seri,

che noi non possiamo più sopportare tutti questi migranti che sbarcano sulle nostre coste. Questo è il messaggio che sta dando il Governo al popolo italiano, non un messaggio di serietà. Peraltro, è un messaggio che è una dichiarazione di impotenza, signora rappresentante del Governo. Con questa legge voi vi dichiarate impotenti, cioè dite di non essere in grado di gestire i flussi migratori, che sono troppo importanti per noi. Ma non fate un accordo per il controllo delle frontiere, perché non mi pare che l'Albania abbia una frontiera con l'Italia. una deportazione in altro Paese, perché non siete in grado di gestire questi flussi in Italia. Le notizie che vengono dai CPR, da tutte le varie situazioni di accoglienza non organizzata, anche in queste settimane, forse dimostrano esattamente questo. Avete alzato le mani, vi siete arresi. Avete detto: non ce la facciamo, ci facciamo aiutare da un Paese che nemmeno ancora aderisce all'Unione europea. Infatti, se questo fosse stato un accordo

al fatto che è una dichiarazione di totale impotenza, essa contiene elementi di incostituzionalità palesi. La prima questione è quella che ha già sollevato, in maniera molto adeguata, il collega De Cristofaro. Come potete scrivere che si applicano, in quanto compatibili, i decreti legislativi relativi all'immigrazione? Questo provvedimento lo abbiamo esaminato in dettaglio in questi giorni e in queste settimane. È un provvedimento caratterizzato da molti condizionali e da molti buchi. Cosa vuol dire che le leggi si applicano in quanto compatibili? Si può applicare una legge in quanto compatibile? Con che cosa? Chi sceglierà i migranti che dalle navi italiane andranno in Albania? Come farete la selezione delle persone? Perché non avete esplicitato i richiami ai decreti legislativi che prevedono che donne in gravidanza, soggetti fragili e minorenni non possono essere oggetto di questa procedura? Perché non è stato esplicitato? Abbiamo presentato emendamenti in tal il primo profilo è che state creando differenze nella selezione delle persone che portate in Albania, in un Paese che non è affatto, come prevede invece la direttiva europea (quindi qui c'è, ancora una volta, una violazione sia costituzionale che dei trattati europei),

è una zona del territorio albanese. Non è una zona di transito di migranti; è una zona di un territorio sovrano e non è nemmeno il territorio di confine. L'altro elemento è: come potete omettere il fatto che le navi italiane sono già territorio italiano? Voi prendete un migrante che, attraverso operazioni di soccorso, viene imbarcato su una nave italiana. Tale nave è già territorio italiano; quindi dal territorio italiano viene portato in territorio albanese, perché non c'è extraterritorialità in quelle aree, e lì si dice che si applica la giurisdizione italiana. Peccato che, per tutte le cose che già sono state dette, il diritto alle informazioni, la consulenza sul diritto di chiedere asilo, il diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza, il diritto di consultare un avvocato o un altro consulente legale ammesso a informare e autorizzato sugli aspetti della domanda di protezione internazionale, tutte queste cose non siano garantite, come invece sono garantite dal diritto UE. Siete stati molto vaghi nel garantire questi diritti, quasi che queste persone fossero oggetto fossero oggetto di una punizione collettiva, di una deportazione collettiva. *(Applausi)*. Cosa penseranno gli altri migranti? Faranno a gara per capire chi è che può rimanere in Italia e chi è che invece viene deportato in Albania. Perché questa differenza? perché il contribuente italiano, invece che chiedere allo Stato italiano di organizzare meglio i suoi *hotspot* e i suoi CPR, dovrebbe essere contento di pagare 600 milioni per per cinque anni per uno o due *hotspot* e un CPR in Albania, quando spendiamo 52 milioni per dieci CPR in Italia? Perché il contribuente italiano dovrebbe pensare che questa sia una soluzione logica, di buona amministrazione, seria, che migliora le condizioni di esame delle domande? Questa dislocazione in Albania complica grandemente tutto: complica l'esame delle domande, complica i diritti del richiedente, complica la gestione delle Forze di polizia, complica la gestione la gestione delle forze della magistratura. Stiamo parlando esattamente di una discriminazione giuridica. Lo straniero portato in Albania, rispetto allo straniero sbarcato in Italia, si troverà in una condizione di discriminazione giuridica, per motivi di condizione personale e non per motivi particolari. Non ha fatto niente di diverso dagli altri, non c'è un criterio di selezione; verrà semplicemente discriminato e avrà meno diritti per una scelta arbitraria, non riconducibile a nessun quadro giuridico serio e quindi in palese violazione del diritto costituzionale.

semplicissima. Quando uno accede alla procedura e richiede la protezione internazionale, non può essere trattenuto negli *hotspot*. In questi *hotspot* albanesi, invece, sarà trattenuto. Il primo ricorso lo perderete,

un messaggio distorto, e cioè che questi migranti, queste persone che vengono a chiedere protezione in Italia devono pagare una pena, devono soffrire di più, devono andare lontani; appena imbarcati, non devono andare nel più vicino posto di sbarco, come prevede la convenzione internazionale *(Applausi)*, devono andare lontani dai nostri occhi, come se lontani dai nostri occhi ci fossero diritti diversi. Se sono lontani dai nostri occhi avranno diritti diversi. Il diritto, la legge dovrebbe rendere chiara a tutti la dignità dell'essere umano e dovrebbe indicare a tutti come questa dignità viene riconosciuta e rispettata.

tutti uguali e di uguale dignità davanti alla legge.

Signora Presidente, quello che preme, credo soprattutto al mio Gruppo, sottolineare e denunciare il furore autoritario che nel metodo ha guidato la gestione di questo provvedimento e il furore ideologico che nel merito lo caratterizza. Oggi

Perché? Forse ci sono delle scadenze improrogabili che vanno rispettate? Forse si tratta di un decreto-legge che prevede una scadenza fissa? No, è un semplice disegno di legge che non ha una scadenza fissa. fissa. È toccato alle opposizioni negoziare in sede di Capigruppo che si potesse tornare in Commissione per provare a finire questo provvedimento. Si è tornati in Commissione, ma non si è conclusa la discussione del provvedimento e ciononostante si arriva in Aula. Si dirà: ci saranno stati migliaia di emendamenti ostruzionistici, per cui ragionevolmente il tempo andava compresso. Presidente, il MoVimento 5 Stelle ha presentato 28 emendamenti. In totale gli emendamenti erano 154. Ora, se le Commissioni riunite affari costituzionali ed esteri non sono in grado di gestire una mole simile di emendamenti - 154 significa o che c'è un'incapacità totale da parte di chi ha il dovere di gestire i lavori *(Applausi)* oppure che non importa la ragionevolezza delle proposte emendative, sia nel merito che nel numero.

tassativamente oggi, tappando quindi la bocca alla critica politica. Quest'ultima ha molto motivo di esserci. Sono state illustrate le pregiudiziali di costituzionalità.

e quindi bisogna portare a punto questo provvedimento iperideologico, che ha un costo

L'elettore di destra dirà che se in tal modo risolviamo l'emergenza immigrazione, come è scritto negli obiettivi tematici di questo provvedimento, sono 650 milioni di euro ben spesi. Ebbene no, Ebbene no, perché con questi 650 milioni di euro il Governo Meloni costruisce due CPR, dove entreranno circa 3.000 persone. Ora, l'elettore di destra, che segue bene il tema dell'immigrazione perché naturalmente ritiene che sia il problema più grande che l'Italia deve affrontare, il suo tallone d'Achille, sa che proprio quest'anno si è toccato il *record* di sbarchi. 150.000! Sotto il Governo Meloni ci

sanità. Si sottraggono quindi servizi essenziali sempre ai contribuenti italiani, tanto per parlare di patrioti, per un investimento assolutamente fallimentare. Con 52 milioni c'è infatti in programma di costruire 10 CPR in Italia. È chiaro allora che qui stiamo parlando di una bandiera propagandistica e ideologica del tutto vuota di contenuti, che rischia però di essere anche incostituzionale. Entriamo infatti nel merito e smettiamola di parlare del vil denaro.

chi è vulnerabile e chi non lo è), vanno in Albania. Quelli invece che a un primo sguardo sembrerebbero vulnerabili possono fare la trafila

illustrate dai miei colleghi De Cristofaro e Delrio. Io ho poche considerazioni da aggiungere per dare conto delle ragioni profonde che ispirano questo voto, ma anche la convinzione delle parole scritte e pronunciate dai nostri colleghi. Intanto una premessa: in quanto a migranti, direi con semplicità che riuscite davvero a superare voi stessi. Avete già varato tanti provvedimenti che io definirei avventati, populistici, ma soprattutto - come veniva ricordato adesso dalla collega Maiorino - inefficaci: dovreste almeno prenderne atto. Questo invece è un provvedimento che, superando anche il decreto Cutro di cui tutti ricordiamo efficacia e conseguenze, riesce addirittura ad essere incomprensibile ai più. Difficile capire i contorni di questo provvedimento e difficile capire come concretamente si realizzerà. Che cosa avete scelto di fare? Sono stati utilizzati anche nella discussione in Commissione termini importanti, che evocano pezzi di storia che vorremmo tutti, convintamente, lasciarci alle nostre spalle che io non ripeterò in quest'Aula, soprattutto per rispetto a quella storia, ma non si può non pensare a quei migranti che vengono soccorsi in mare in condizioni che spesso rasentano la sopravvivenza e invece di portarli - come disciplinano i diritti internazionali e il diritto del mare - nel porto più vicino e più sicuro, li li mettiamo su una nave, che è territorio italiano, e facciamo fare loro altri due giorni di viaggio per non sapere bene dove li porteremo, in un contesto che non abbiamo capito se è disciplinato dalle leggi italiane, se sia territorio italiano, che strutture siano, che personale ci sarà, che livello di accoglienza, che livello di intermediazione,

e umanamente comprensibile, anche se ingiustificabile. Il tema vero è che potete porvi in una logica di maggioranza e di prove di forza, ma non vi potete ancora porre al di sopra della Costituzione. Allora, quando scrivete nei vostri provvedimenti alcuni riferimenti normativi, quando questi provvedimenti dovranno essere concretamente adottati e applicati da un giudice di fronte a una controversia - e da questo provvedimento scaturiranno controversie, perché è veramente di difficile interpretazione, ma soprattutto applicazione ebbene quel giudice si rivolgerà alla Corte. Questo provvedimento non potrà mai superare il vaglio della Corte nel momento in cui scrive che queste norme si applicano «in quanto compatibili», perché l'articolo 117 della nostra Costituzione è chiaro e dice che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Non scrive «in quanto compatibili»

sarà un atteggiamento che voi provate a perorare, ma che di fronte a un giudice della Corte costituzionale con ogni evidenza non reggerà. Quindi, la vostra propaganda, il vostro populismo, giocato ancora sulla pelle dei più fragili e dei più esposti, non vi ripagherà e gli italiani saranno accorti, ma forse anche i giudici saranno più severi, nel dirvi che non solo impegnate risorse importanti di questa legge di bilancio in un tempo nel quale le risorse sono preziose, ma che avremmo potuto utilizzarle probabilmente per migliorare per migliorare il sistema di accoglienza che voi continuate a debellare *(Applausi)* e che è l'unica vera arma che abbiamo per tentare di fare di questi migranti persone con dignità. È l'unica vera strada maestra che abbiamo per garantire maggiore sicurezza nel nostro territorio, perché integrazione e sicurezza camminano insieme, non certo mortificazione e umiliazione e soprattutto un atteggiamento - come veniva ricordato prima - punitivo e discriminatorio nei confronti delle persone. Quelle messe ai margini sociali saranno sempre e per forza persone più insicure: questo lo ricordo anche alla becera propaganda fatta fatta qualche giorno fa rispetto alle vicende drammatiche di Catania. È la marginalità sociale che rende insicuro il nostro Paese *(Applausi)*, non la provenienza delle persone:

esserlo, come abbiamo detto in Commissione, e non solo il tema del garantismo e delle garanzie costituzionali previste dal diritto di difesa, richiamate dalla pregiudiziale del collega De Cristofaro con riferimento all'articolo 24 della nostra Costituzione. L'articolo 3 - lo ribadisco - dice che tutti abbiamo pari dignità, siamo uguali; di fronte al nostro Stato e alle leggi del nostro Stato siamo uguali. Che si venga via mare o via terra, siamo uguali. *(Applausi)*. Non si giustificherà perché alcuni verranno portati in luoghi che saranno necessariamente difficili, più complicati, dove l'intermediazione culturale sarà sicuramente più difficile, dove il diritto di difesa sarà più difficile, dove la loro qualità della vita sarà messa a dura prova. Viene messa a dura prova anche per i migranti in Italia, ma è evidente che un centro costruito

dividerete o qualificherete una madre incinta che viene divisa dal suo compagno o da un altro figlio? *(Applausi)*. Diteci in virtù di quale valutazione dividerete famiglie, genitori, mamme, bambini; alcuni li manderete in Albania e altri li manderete qui in Italia, Con quale coraggio una mamma la dividete da un bambino di quattro o cinque anni? Come fate a qualificare una donna vittima di violenza? Ne abbiamo parlato anche in occasione del cosiddetto decreto-legge Cutro. Abbiamo detto che una donna vittima di violenza che intraprende un viaggio probabilmente ha subito quella violenza durante il viaggio; non ne è nemmeno consapevole in alcuni casi o è addirittura accompagnata dalla persona che le ha esercitato violenza. Vi avevamo chiesto di introdurre nei centri di accoglienza qui in Italia personale ed operatori specializzati. Non lo avete fatto, non lo avete messo lì e adesso pensate che andiamo sulle navi e distinguiamo distinguiamo le persone vulnerabili da quelle non vulnerabili, portiamo personale specializzato, riusciamo a definire le persone che sono vulnerabili e quelle che non lo sono e a quel punto dividiamo? Dividiamo quelli che per voi sono carichi residuali, mentre per noi sono persone piene di dignità *(Applausi)*, che meritano rispetto e assistenza, e sulle quali la nostra scommessa è solo una: integrazione e dignità.

il piano Mattei e il Protocollo che stiamo discutendo oggi sono figli di un'unica visione che vede il problema immigratorio al centro e sono tasselli di un unico mosaico che stiamo ricomponendo pian piano in questi lunghi mesi. parte dimostrano che le norme, per trovare la loro efficacia, hanno bisogno di tempo: di mesi e a volte anche di anni. Se prendiamo i dati del Viminale da ottobre ad oggi, ci rendiamo conto che i flussi migratori sono diminuiti del 30 per cento, con picchi anche del 50 per cento. Quando quest'ultimo provvedimento avrà piena efficacia i dati scenderanno ancora, con buona pace dei detrattori del Protocollo in esame. È un provvedimento che mira alla cooperazione, non certo a un'imposizione, che esclude, nel pieno rispetto del diritto internazionale, i minori, le persone vulnerabili, le donne in gravidanza e questo con buona pace

È un provvedimento complesso che, però, mira anche all'organizzazione precisa degli *hub* sul territorio albanese e crea due aree: una portuale, l'altra più interna, sulla quale verranno destinati i migranti. Saranno delle vere e proprie aree a controllo italiano al loro interno; nella parte esterna, invece, la potestà rimarrà di competenza delle Forze di polizia e delle autorità albanesi.

il fatto è che oggi noi cerchiamo di risolvere un problema che in più di dieci anni non siete riusciti a risolvere. Lo facciamo anche con spirito di solidarietà, la verità è che voi siete i soliti antitaliani *(Applausi)*, per cui qualsiasi cosa si faccia a favore dell'Italia, se ciò porta beneficio all'Italia e all'operato del suo Governo, vi vede contrari.

il presidente Rama ha accettato la richiesta di cooperazione avanzata dall'Italia? È una domanda che io mi sono posto. Lo ha fatto per uno spirito di riconoscenza, perché nel 1991, quando i cittadini albanesi si ribellarono al regime comunista albanese, il primo Paese che accolse gli albanesi fu l'Italia *(Applausi)* e ci sta facendo tornare indietro solo quella solidarietà che noi mostrammo trent'anni fa. Mi rendo conto che questo per voi sia un pugno nello stomaco difficile da digerire, perché quando anche questo provvedimento avrà piena efficacia, l'afflato tra il Governo italiano e i cittadini italiani sarà ancora maggiore.

hanno più volte detto che prenderanno addirittura a modello questo trattato vuol dire che siamo sulla strada giusta. Venendo alla sostanza del problema, il trattato è stato definito inquietante, pericoloso, illegale, contrario al senso di umanità, illegittimo e inefficace. Invece sarà un modello, sarà un vero e proprio deterrente che disincentiverà la migrazione economica; sarà un duro colpo per i mercenari della clandestinità adorata, per gli approfittatori, per gli scafisti, per tutte le organizzazioni criminali che, con questo *humus* marcio, lucrano e si alimentano Sarà un duro colpo anche per i vostri amici delle ONG, che spesso e volentieri violano il diritto italiano *(Applausi)*. Servirà anche ad altro, perché ci farà comprendere davvero chi scappa perché fugge da una guerra e dalla fame e chi, invece, quel diritto non ce l'ha. ce l'ha. Chi scappa da guerra e fame, infatti, non si pone il problema di dove arriva; chi scappa da guerra e fame si pone il problema di dove sta e da lì vuole scappare. Chi si pone il problema di dove vuole arrivare, invece, dovrà sapere che da oggi in poi può arrivare anche in Albania, non per forza in Italia. Papa Benedetto XVI affermava che il primo diritto di un migrante è quello a non emigrare e lo diceva seguendo le parole di un altro grande Papa, Giovanni Paolo II, che nella sua enciclica «*Ecclesia in Europa*» affermò che la Chiesa ha il dovere dell'accoglienza, ma è responsabilità delle autorità pubbliche esercitare il controllo dei flussi migratori nel rispetto delle leggi e quindi coniugarsi, quando necessario, con la ferma repressione degli abusi. Ecco, è in quella direzione che sta andando il Governo italiano e lo sta facendo nel pieno rispetto del diritto interno e del diritto internazionale, perché è bene che su questo principio ci ritroviamo tutti quanti: la difesa dei confini è un diritto sacrosanto, non è un'opzione esercitabile a seconda dei casi.

è difficile anche entrare nel dettaglio di questo provvedimento, perché è talmente scombiccherato, illogico, irrazionale

razionale che può aver indotto il Governo italiano a chiedere al Governo albanese di prestarsi a quest'obbrobrio, a questa specie di mostro

di mostro giuridico, a questo bizzarro accordo internazionale sono i numeri, perché, come si diceva già in precedenza, nel 2023 sono sbarcati in Italia 155.754 migranti,

di quelli sbarcati nel 2021 (67.040). Signor Presidente, ho avuto l'onore e la ventura di servire al Governo della Repubblica proprio al Ministero dell'interno e di essere stato Sottosegretario di una servitrice dello Stato, una professionista al cui rigore professionale dovremmo inchinarci, che risponde al nome di Luciana Lamorgese, che è stata messa in croce con un tiro al bersaglio quotidiano da parte di una maggioranza che le imputava qualsiasi cosa succedesse nel Paese. Ebbene, mi chiedo che cosa direbbero oggi Fratelli d'Italia e la Lega se al Viminale ci fosse Luciana Lamorgese. Il silenzio che invece giunge dai banchi alla mia sinistra e alla sua destra, signora Presidente, è segno di un chiaro imbarazzo. Voglio ricordare a tutti

«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica» - non all'estero - «secondo le condizioni stabilite dalla legge». Quello che sta succedendo qui è esattamente la negazione non tanto della lettera, ma dello spirito della nostra Costituzione, che riconosce universalmente a tutti gli esseri umani dignità, il diritto di realizzazione della propria personalità, la protezione nel momento della difficoltà e appunto il godimento di quei diritti democratici che stanno scritti nella Costituzione. Il pensiero che persone che arrivano sul nostro territorio nazionale vengano trattate alla stregua dei rifiuti che mandiamo nei Paesi stranieri perché non sappiamo cosa farcene, che è quello che succede in Italia con i rifiuti veri e propri, che vengono caricati su treni e camion per essere smaltiti altrove, è un'immagine che credo

questo non è chiaro, quindi certamente ben prima della Corte costituzionale sarà la realtà a dire che questa costruzione, fragilissima e ideologica, collasserà su se stessa. Ciò che è più grave, però, è che non comprendete che in questo Paese c'è una drammatica crisi demografica, che non risolveremo certamente solo

per comprendere come trasformare l'immigrazione in una risorsa per un Paese che ha un disperato bisogno di braccia e cervelli, pensate a questi meccanismi di discarica all'estero, vuol dire che non avete capito niente. Scusate la franchezza, cari colleghi, ma non avete capito che qui andremo a chiudere gli gli ospedali e che non avremo insegnanti per i nostri bambini. Allora, invece di tirar fuori ridicoli conigli dal cilindro, per favore, mettete via l'ideologia e provate, pragmaticamente, a risolvere i problemi del Paese.

A me sembra che, probabilmente, questa sia l'ultima spiaggia per un Governo che, fino ad oggi, ha adottato soltanto politiche fallimentari. Diciamocelo chiaramente: avete iniziato con un decreto sulle ONG, che non ha prodotto effetti. Avete proseguito con il decreto Cutro uno, con il decreto Cutro tutti decreti-legge che non hanno modificato il problema. Questo perché? Perché non siete stati in grado di agire sulle cause e state agendo soltanto sugli effetti. *(Applausi)*. A me sembra che vi stiate cimentando in un eterno gioco dell'oca, dove ogni nuovo passo avanti è sempre un ritorno al punto di partenza, però, in questo vostro gioco, il problema è che sembra siano stati accantonati i diritti umani e che la dimensione umana di un problema epocale sia passata in secondo piano. E questo è terribile, perché state mettendo in secondo piano i diritti dei migranti per dare spazio a una retorica dell'odio, dei respingimenti e dei blocchi navali.

distorta attraverso la lente della vostra indifferenza e dell'insensibilità verso i diritti delle persone. Cerchiamo di essere chiari: questo provvedimento non risolve il problema. È semplicemente un modo per nascondere la realtà sotto al tappeto, come facevamo all'università, quando non volevamo dimostrare alla mamma di non essere in grado di tenere la cameretta in ordine, allora nascondevamo le cose sotto il letto; non risolve il problema, crea soltanto un'illusione: date agli italiani l'illusione che il problema non esista, semplicemente perché non lo rendete visibile; però, vedete, questa illusione costa agli italiani quasi 700 milioni di euro. Sia ben chiaro, Presidente, il Governo è libero di decidere come spendere i soldi degli italiani; però poi non venite a raccontarci la storia della coperta corta. corta. Non ci potete dire che non ci sono i soldi per realizzare le infrastrutture e bocciate gli emendamenti sull'autonomia differenziata; non ci potete dire che non ci sono soldi per la sanità e che non ci sono soldi per creare sviluppo nelle aree di crisi industriale complessa. C'è un altro paradosso in questa vostra politica sull'immigrazione. Adesso addirittura vi volete dipingere come i benefattori del continente africano e dite che, attraverso il Piano Mattei, volete creare le basi per lo sviluppo del continente africano. Ma se non siete stati in grado di creare sviluppo neppure in Italia, come pensate di risollevare le sorti del continente africano? Cercate di essere onesti e ammettetelo: avevate detto di essere pronti a governare, ma avete dimostrato di non esserlo. Abbandoniamo questa retorica del nulla: è venuto il momento in cui ci dovete dimostrare non di essere pronti a governare, ma di essere in grado di farlo.

Ragazzi, ma se volete riconoscere questo diritto a non emigrare, l'unica politica che dovete fare è quella della cooperazione internazionale. Questa gente non viene qui soltanto per divertimento. Dovete creare le condizioni, nei Paesi d'origine, affinché le persone non debbano scappare perché non ci sono gli ospedali e si rischia di morire per la puntura di una zanzara, perché non sanno dove mandare i figli a scuola i figli a scuola o perché ci sono le guerre. Dovete fare opere di diplomazia e non politiche di natura belligerante, come state mostrando di fare. Colleghi, qui però c'è davvero bisogno di un cambio di prospettiva. Andiamo alla base e concludo, Presidente. Qui il problema e la vera minaccia non sono quello che si teme; la vera minaccia sono le conseguenze a cui può portare questa costante paura di essere in pericolo. Vorrei ricordare, Presidente, che i totalitarismi sono nati proprio su questa paura e su questa esigenza di ordine e disciplina, perché si sono proposti come in grado Le lascio un minuto, però i tempi sono contingentati. si intitolava "Come si diventa nazisti". Il particolare di questo saggio è che narra di un piccolo paesino di gente perbene. L'unica loro caratteristica era la paura verso un presunto nemico, magari all'epoca erano gli ebrei. ebrei. Su questa base di paura e su questo bisogno di ordine e disciplina si è aperta la strada ai nazisti, che si sono proposti come i distributori di sicurezza e di certezza e coloro che potevano dare maggiore tranquillità al cittadino perbene.

ci accingiamo a votare un provvedimento che non solo costerà molti soldi ai contribuenti italiani, ma che soprattutto non servirà a risolvere la gestione dell'immigrazione irregolare in Italia. Prima ancora di vedere perché non serve, consentitemi di richiamare la vostra attenzione su un dato: il Senato oggi, e prima la Camera, sta discutendo di una questione rilevante per il nostro Paese e lo sta facendo solo grazie all'insistenza

Invece siamo qui a discutere e, dopo aver approfondito ulteriormente le norme contenute in questo Protocollo, siamo sempre più convinti che sia solo l'ennesimo atto di distrazione di massa del Governo Meloni sul tema dell'immigrazione. Dopo i fantomatici blocchi navali e i porti chiusi, oggi si contano - come ha già ben ricordato il collega Scalfarotto - oltre 150.000 ingressi, a sancire un fallimento clamoroso delle vostre politiche migratorie. Nonostante questo, si continua a perseverare ora con tale accordo truffa con l'Albania, perché non sapete nemmeno voi cosa ci andiamo a fare nei centri, in Albania. e non è una questione di lana caprina - nessuno sa dove saranno identificati i migranti, se in Albania o a bordo delle navi che hanno effettuato il soccorso - è una questione mai chiarita tenendo presente che generalmente non hanno carta d'identità o passaporto e per scoprirlo servono persone adatte con strumenti adeguati, come la conoscenza delle lingue; poi servono anche le autorità consolari che confermino la loro nazionalità. Insomma, è un lavoro complesso e costoso che ancora adesso non sappiamo esattamente come si intenda svolgere. Nessuno sa bene con esattezza come ci si debba comportare con un minore non accompagnato, con un disabile o con gli anziani (e chi stabilisce quando si è anziani?). Poi ci sono persone che hanno subito torture, stupri e violenze, le vittime di tratta, i nuovi nati, come precisa il testo del Protocollo. Insomma, è davvero complicato capire come saranno identificate identificate queste persone, anche perché il personale delle navi non ha queste competenze e, di conseguenza, quello che auspicate non è percorribile. Insomma, non riusciamo davvero a comprendere che senso abbia realizzare un centro in Albania che dovrà ospitare non più di 3.000 persone, anziché

tutta propagandistica, di dimostrare che siamo efficienti, capaci di tenere lontani dalle nostre spiagge gli immigrati? O forse, più prosaicamente, perché, nonostante le dichiarazioni di governatori e sindaci di destra, quei centri nessuno li vuole vicino a casa. Ricordate? Il ministro Piantedosi ci aveva detto che avrebbero fatto un *hotspot* per Regione, anche due: altri annunci, parole al vento. Noi quindi spenderemo più o meno 700 milioni in pochi anni per 3.000 persone, ma vorrei ricordare che a Trieste, attraverso la rotta balcanica, in pochi mesi sono arrivate 14.000 persone, molti minori, diversi dei quali non accompagnati, costretti a vivere per strada, nei silos, un vecchio edificio veramente in disuso, tra topi e serpenti. Per questo non si trovano finanziamenti. Nulla: una vergogna! Lo straniero portato in Albania rispetto a quello sbarcato in Italia si troverà in una condizione di discriminazione giuridica per motivi di condizione personale espressamente vietata anche dalla nostra Costituzione. Sono allarmanti inoltre gli oneri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato, che l'Italia dovrà sborsare

risorse sottratte alla sanità, all'istruzione, alla cultura, ma soprattutto non date ai Comuni per le politiche di accoglienza, che servirebbero in questa situazione.

siamo chiamati a discutere la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra il Governo italiano e quello albanese in materia migratoria, un accordo che introduce una modalità sicuramente innovativa nella gestione dei flussi migratori, della quale è presupposto la consolidata e storica amicizia fra l'Italia e l'Albania. Questo provvedimento non è uno *spot* o un'iniziativa isolata, ma rientra in una visione strategica della questione migratoria e in un posizionamento molto attento dell'Italia, che acquisisce nuova centralità nello scenario internazionale, due temi e due aspetti che sono sicuramente collegati. Abbiamo infatti dati molto incoraggianti da questo punto di vista: mediamente, un 30 per cento in meno di sbarchi. Non è il nostro approdo finale, ma è un obiettivo importante, frutto di una politica attenta e programmata. Ci sono risultati importanti che aumentano la credibilità dell'Italia e ci consentono di portare avanti questa strategia, che sono visibili in tutti gli elementi della nostra politica internazionale, nella centralità nelle politiche europee, nella capacità di influire sui *dossier* principali. Potremmo parlare anche della direttiva sui pesticidi o di quella o di quella sugli imballaggi e di come l'Italia sia stata determinante nel cambiare l'approccio dell'Europa su quei temi e, naturalmente, anche su quello migratorio. a un anno fa, prima dell'avvento del Governo di Giorgia Meloni, alcune delle parole che oggi sono pienamente nell'agenda dell'Unione europea erano impronunciabili. Semplicemente e banalmente non si poteva di difesa dei confini nazionali ed europei. Abbiamo introdotto questi temi nell'agenda europea e abbiamo affrontato a 360 gradi il fenomeno migratorio, mettendo in campo iniziative di deterrenza e di contrasto all'immigrazione illegale, sostenendo allo stesso tempo, presupposto per quest'apertura, il contrasto fermo all'immigrazione illegale aprendo invece ai flussi migratori controllati, dei quali in una modalità organizzata, attenta e studiata abbiamo anche bisogno. Da questo punto di vista, contrastare l'immigrazione illegale significa salvare vite e, come abbiamo fatto con il cosiddetto decreto Cutro, inasprire

internazionali sul tema dei rifugiati e sul tema di coloro che scappano dai conflitti. Rispetto però a un tema macroscopico come quello di un'immigrazione di massa legata ai temi economici, al cambiamento climatico e alla povertà, serve altro rispetto a quello che abbiamo ascoltato anche oggi da parte delle opposizioni ovvero una politica che non si capisce poi quale dovrebbe essere, se non sicuramente non attenta al controllo dei confini.

e delegazioni dell'Africa erano qui a parlare di azioni proattive che dobbiamo fare. Voi amate difendere il diritto ad emigrare, noi vogliamo invece difendere il diritto a non emigrare di quei popoli *(Applausi)*, a una cooperazione che non sia predatoria da parte dell'Occidente, ma che sia paritaria e che può essere una grande operazione di mutuo soccorso per noi e per quei popoli. È stato anche importante vedere l'Europa accogliere questa iniziativa dell'Italia e quindi, per una volta, diversamente da quello che avveniva con i Governi precedenti, non l'Italia acriticamente dietro all'Europa, ma l'Europa costruttivamente dietro e a fianco dell'Italia.

e nuovi CPR per il collocamento temporaneo dei migranti tratti in salvo dalle nostre autorità. Voglio dire, da questo punto di vista, che lascia un po' basiti il tentativo di screditare questo accordo, che poi diventa anche un tentativo di screditare

vergognosi attacchi subiti in questi giorni. *(Applausi)*. Avete dimostrato anche un certo attaccamento a quello strumento di lancio tipico degli aborigeni australiani che è il *boomerang*, perché avete

il testo di cui discutiamo oggi, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, mi costringe a fare un doveroso passo indietro e ricordare come siamo arrivati a questo punto. Ebbene, erano i primi di novembre del 2023, quando la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, annunciò alla stampa, non al Parlamento, di aver sottoscritto un Protocollo con il Presidente dell'Albania per la gestione degli immigrati irregolari. Lo stupore fu notevole, non soltanto per il tema del Protocollo, ma anche e soprattutto perché il Parlamento ne veniva informato a mezzo stampa. Prima non se ne era parlato, non si conosceva neanche il testo, né di cosa parlasse esattamente, tanto che i dettagli vennero poi forniti dai Ministri del Governo. Addirittura il ministro Fitto disse testualmente: «per la prima volta uno Stato non membro dell'Unione europea, ancorché candidato, accetta la creazione sul suo territorio di centri destinati alla gestione dei migranti illegali arrivati sul territorio dell'Unione».

coacervo di norme messo in piedi dal Governo, che pone numerosi quesiti di legittimità costituzionale, che non ho dubbi verranno sollevati e risolti nel senso peggiore possibile, cioè con un vaglio di costituzionalità che non verrà superato per una serie di ragioni: non perché siamo antitaliani, ma, al contrario, siamo così tanto italiani da volere che il legislatore legiferi bene e sapendo di farlo in conformità con la Costituzione. E quando ha un dubbio sulla legittimità della Costituzione - e qua di dubbi, oggettivamente, ce ne sono tanti - si fermi e riveda quello che vuole fare. Infatti, non è corretto promulgare una legge quando già si sa che è affetta da numerosi vizi. Il primo di questi è l'extraterritorialità. Sarà difficile, Presidente, in sei minuti dire tutto quello che vorrei dire, perciò stringerò, condenserò e cercherò di dire le cose essenziali. Il primo vizio è l'extraterritorialità, come abbiamo detto anche nella questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. Come si può Come si può pensare di realizzare un centro per la gestione dei migranti irregolari nel territorio di uno Stato estero che non fa neppure parte dell'Unione europea? questione abnorme dal punto di vista giuridico: "abnorme" in senso letterale, cioè noi andiamo oltre le norme, oltre le disposizioni vigenti. Lo spiego in termini chiarissimi e semplicissimi: la legislazione italiana ovviamente riconosce quella europea come fonte sovraordinata. La legislazione albanese ovviamente no, per la semplice ragione che non fa parte dell'Unione europea. Noi creiamo un centro sul territorio albanese, all'interno del quale mettiamo i migranti che siamo andati a prevelare in mezzo al mare nelle acque territoriali, stabilendo che non li porteremo nel centro di primo soccorso, come sarebbe più facile, ma direttamente in Albania e in quella sede, quando li sbarcheremo, diremo loro che saranno sottoposti alla legislazione italiana. Presidente, immagino che lei mi potrebbe dire: in quel centro si applica il principio di extraterritorialità e vale la legge italiana per tutti. Io le risponderei di no: al contrario, in quel centro si continua ad applicare la legge albanese, perché si trova sul territorio albanese; solo per i migranti italiani si applicheranno le disposizioni della legge nazionale italiana e di quella comunitaria. Questo crea un incidente e una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del diritto di difesa. Sono questioni abnormi, per per la semplice ragione che lo stesso Protocollo, all'atto pratico, chiarisce: se dentro questi centri venisse commesso un delitto, una rissa o un furto,

un migrante, allora sarà sottoposto alla giurisdizione della legge italiana e alla legislazione italiana, cioè applicheremo la legge italiana. Se però il migrante dovesse compiere un delitto nei confronti di un cittadino albanese o dello Stato albanese, allora si applicherà la legge albanese.

che il migrante nel procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato verrà sentito in videocollegamento con un avvocato che non avrà neanche modo di ascoltarlo personalmente, è una violazione del diritto di difesa sostanziale e comporterà la condanna dell'Italia per la violazione dei diritti umani e dei diritti di difesa dei migranti. Perché facciamo questo Protocollo con quest'urgenza e con questa fretta? Non è stato consentito neanche alla 1a e alla 3a Commissione riunite di completare l'esame e la discussione degli emendamenti. Per quale motivo? Quale urgenza c'è? Non c'era alcuna urgenza, anche perché questa misura è inadeguata a risolvere il problema della migrazione, non soltanto per le evidenti violazioni dei diritti comunitari e della dignità delle persone, ma anche dal punto di vista numerico. Questo centro Questo centro accoglierà al massimo 3.000 persone. La quota dei migranti arrivata in Italia nel 2023 è 157.000, il che significa che soltanto una piccolissima parte di essi potrà essere accolta nel centro in Albania. A fronte di questo sforzo

non ci siano motivi razionali, dal punto di vista della legge e neanche dell'opportunità per procedere alla ratifica di questo Protocollo. Ci sono soltanto motivi di propaganda politica

Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, come sappiamo, è rimasto per settimane molto opaco. All'inizio, il Governo addirittura pensava di affrontare questo tema senza passare dal Parlamento; poi forse ha letto la Costituzione e quindi ha dovuto farlo. Non ho la soluzione in tasca per affrontare e risolvere i problemi dell'emigrazione, però è chiaro che quello che qui viene proposto è un percorso

cercando di non farle vedere. Il problema è che gli immigrati, in particolare quelli che arrivano dal mare, hanno un colore scuro e quindi si vedono in qualsiasi posto li mettiamo.

Inoltre, parliamoci chiaro: l'emigrazione è dipesa anche dalla rapina che l'Occidente ha fatto in molti Paesi, a partire dall'Africa, ma non solo. Io seguo la questione da molti anni e vado nei campi profughi, ad esempio della rotta balcanica; andare a vedere quando arrivano i ragazzi che nella loro vita hanno visto solo guerra, ad esempio gli afgani; vi invito a vedere cosa hanno combinato prima i sovietici e poi gli americani, cioè prima l'Oriente e poi l'Occidente.

li prendiamo a legnate e li mandiamo indietro. Questo è il modello che è stato applicato in tutti questi anni sulla questione dell'immigrazione. Come ho detto prima, non ho la soluzione, perché è un tema complesso, però forse bisogna cambiare radicalmente l'impostazione. Il problema è che ci sono migranti economici perché nel loro Paese la situazione è disastrosa, magari,

ho presentato un'interrogazione in cui chiedo la chiusura dei CPR, perché sono *lager*

Uso un termine forte, perché quando vedete le foto di cos'è successo nel CPR di via Corelli vi viene la pelle d'oca. Anzi, è difficile discutere dal punto di vista politico: io sto male, quando vedo quelle foto. Basta pubblicarle, queste foto,

persone vengono messe in un posto in cui la giurisdizione è tutta italiana e non hanno neanche la possibilità di avere vicino i parlamentari del nostro Paese che possano visitarli, o che gli avvocati siano vicini, vengono meno i loro

Il 23 marzo 2023 c'è lo storico cambio di passo in Europa grazie a Giorgia Meloni e il tema dei migranti diventa centrale al Consiglio europeo. Sì, così centrale da meritarsi due righe in fondo al protocollo in cui è scritto che se ne parlerà a giugno. L'8 giugno 2023 c'è l'accordo storico sul nuovo patto sui migranti, sempre targato Giorgia Meloni, naturalmente. Peccato che non ci sia stato alcun sostanziale cambiamento perché l'Italia resta il Paese che dovrà occuparsi da solo da solo di arrivo, accoglienza e gestione dei migranti, esattamente come prima, senza alcun obbligo di redistribuzione; obbligo a cui si è strenuamente opposto l'amico Orbàn, che la patriota Giorgia Meloni ha ben compreso, perché per l'Ungheria si trattava di difendere i propri interessi nazionali, con buona pace degli interessi nazionali degli italiani, naturalmente. 17 luglio 2023 c'è la storica intesa con la Tunisia. Si tratta forse di un duro colpo ai trafficanti di vite umane che da questo momento in poi non riusciranno più a partire dalle coste tunisine? Un nuovo colpo per i trafficanti che, dopo il decreto Cutro, già avevano il loro bel da fare a scappare inseguiti dalle autorità italiane per tutto il globo terracqueo? Certamente no, perché vengono messi solo pochi spiccioli per i controlli delle frontiere e non viene fatto niente nemmeno sul piano dei rimpatri, perché riguardano solo i migranti tunisini che rappresentano una percentuale infima rispetto ai migranti subsahariani.

continuando con questo ritmo di quattro svolte storiche all'anno, i libri di storia contemporanea dovranno dedicare un volume a parte alle gesta della presidente Meloni. *(Applausi)*. Ma fuori dalla propaganda, nella realtà dei fatti, l'unica svolta storica è il *record* di sbarchi del 2023: 157.000 migranti arrivati in Italia, un rotondo più 50 per cento contro cui si è infranta tutta la vostra vuota retorica. Nella realtà dei fatti c'è la Giorgia Meloni che, al telefono con due comici russi, pensando di parlare con il presidente della Commissione africana Moussa africana Moussa Faki, ammette che sul tema migranti, quando chiama gli altri *leader* europei, non le rispondono nemmeno al telefono. il vero Moussa Faki, lo scorso 29 gennaio, ha smascherato l'ennesimo *bluff* spacciato per atto storico di questo Governo, il Piano Mattei. Il presidente Moussa Faki, infatti, ha dichiarato che l'Unione africana non era stata nemmeno consultata: alla faccia del partenariato paritario! E ha proseguito che non bastano le parole e le promesse, ma servono i fatti. Passiamo ai fatti, ai numeri di questo Protocollo tutto fuffa e propaganda: 650 milioni di euro sarà il costo che sosterrà l'Italia in cinque anni per portare in Albania i migranti sbarcati sulle coste italiane; circa 3.000 saranno i migranti che potranno essere ospitati nella struttura albanese. Diciotto mesi dopo il trasferimento, i migranti non rimpatriati, praticamente il 90 per cento in base alle ultime statistiche, torneranno in Italia. Cosa ci dicono, allora, questi numeri? Ci dicono che gli italiani pagheranno di tasca propria la campagna elettorale di Giorgia Meloni per le prossime europee, sborsando circa sette volte il costo di una struttura equivalente sul territorio italiano. Ma come? La Meloni non ha fatto un'intera campagna elettorale attaccando le misure di dignità, come il reddito di cittadinanza, e di rilancio dell'economia, come il superbonus, dicendo che erano soldi buttati dalla finestra per raccattare voti? Ma questi sapete come li definirebbe la Giorgia Meloni dell'opposizione? Soldi degli italiani, del sangue Questi numeri ci dicono che non ci sarà nessun tangibile risultato nell'alleggerimento della pressione sulle coste italiane, perché i migranti trasferiti in Albania non arriveranno nemmeno al 2 rispetto ai numeri registrati nel 2023. Infine, la cosa più preoccupante è che questo Governo dimostra di non avere la minima idea di come gestire *dossier* così pericolosi, visto che eravate pronti a gestirli,

riconoscenza nei confronti dell'Italia per quello che è stato fatto. Intervistato, Edi Rama ha candidamente detto che Giorgia Meloni si è rivolta a lui perché è frustrata. Secondo lei, l'Unione europea non considera l'immigrazione un problema comunitario. Allora, speriamo davvero che quel telefono, cui non hanno risposto gli altri *leader* europei, smetta di squillare a vuoto, perché sedare la frustrazione del presidente Meloni con questo Protocollo costerà 650 milioni di soldi degli italiani.

Quello che differenzia destra e sinistra è, invece, l'approccio politico da attuare per la gestione di questa problematica, che negli ultimi decenni ha assunto le dimensioni che tutti noi oggi conosciamo. Sul tema, per noi della Lega l'immigrazione irregolare incontrollata è illegale, non è mai stata tollerabile e continua a non esserlo. Spesso, in nome di un approccio ideologico di accoglienza indiscriminata, si sono create le condizioni di pericolo sociale, di insicurezza e, a volte, anche di rischio terroristico per l'Italia e i vari Paesi europei; ideologia che, direttamente o indirettamente, ha creato una cortina fumogena dietro la quale si sono celati, e a volte protetti, interessi economici e *business* criminali e si sono nel contempo - male nel male - tradite le legittime attese di chi vuole diventare cittadino italiano seguendo le procedure previste, nel pieno rispetto delle leggi e delle consuetudini del nostro Paese. Solo uno Stato che sappia difendere con fermezza e convinzione i propri confini è in grado di garantire l'inserimento e l'integrazione nella comunità nazionale di nuovi cittadini. Come dicevo, da sempre questo principio guida l'azione della Lega. Il nostro segretario Matteo Salvini, da Ministro dell'interno, è stato investito nel 2018 di un preciso mandato popolare, che lui ha coraggiosamente rispettato: fermare gli sbarchi. E così è stato. dei nostri confini ha sortito l'effetto di annullare quasi completamente gli sbarchi illegali, riducendo drasticamente le morti in mare e salvando la vita di tante persone cadute nelle mani di scafisti senza scrupoli. I numeri parlano chiaro: nell'anno di Salvini come Ministro dell'interno abbiamo avuto meno 80 per cento di immigrati sbarcati, meno 55 per cento di presunti dispersi in mare, cento di cadaveri recuperati in mare. Questi sono fatti, il resto sono chiacchiere. possiamo dire orgogliosamente agli italiani che sul tema dell'immigrazione Salvini e la Lega hanno la coscienza a posto e le carte in regola. Salvini ha attuato quello che aveva promesso agli italiani e che - aggiungo, Presidente - è stato messo nero su bianco nel contratto di Governo e aveva il pieno sostegno dell'intera maggioranza, compreso il MoVimento 5 Stelle, i cui esponenti, che oggi ci fanno la lezioncina, allora facevano a gara a intestarsi i successi di Salvini. Conte dagli Stati Uniti dichiarava, intervistato da Fox News che, da quando il suo Governo si era insediato, l'immigrazione illegale era crollata in modo ingente, e parlava dell'80-85 per cento in meno rispetto all'anno

ma Salvini con lui e con il presidente Conte, avevano diminuito di una cifra davvero enorme il numero degli sbarchi. Significava che stavano facendo un buon lavoro di squadra. Quella squadra, che allora si vantava dei risultati di Salvini, con un vergognoso voltafaccia ha cambiato rapidamente idea *(Applausi)* e, per fare un Governo con la sinistra che sosteneva l'opposto, ha cancellato i decreti Salvini e, con un voto vergognoso, ha trasformato una linea politica in un fatto giudiziario. E Salvini oggi è a processo con l'accusa ridicola di sequestro di persona. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Un voto inaccettabile e aggiungo anche miope politicamente, che direttamente o indirettamente - non nascondiamoci - è stato uno dei fattori del ritorno ad una degenerazione dei numeri relativi agli sbarchi. è stato accompagnato da un'integrazione dei nuovi arrivati che è sempre difficile e spesso impossibile, per diversità culturali insormontabili ed episodi di delinquenza di cui si rendono quotidianamente protagonisti immigrati sbarcati illegalmente sulle nostre coste. L'esperienza pertanto ci mostra qual è la via maestra da seguire: fermezza nel blocco degli ingressi, a cui è ovviamente opportuno accompagnare una politica di collaborazione e partenariato a diversi livelli con altri Paesi del Mediterraneo. L'accordo con l'Albania va in questa direzione. La ratifica ed esecuzione del Protocollo è un ritorno alla politica del fare che non aspetta gli eventi o invoca l'intervento di un'Europa perennemente assente. È un accordo bilaterale che rappresenta una forma sperimentale di creazione di *hotspot* fuori dal territorio nazionale, ma gestiti dall'Italia secondo le leggi italiane, che la Lega appoggia. Intanto, purtroppo la vita reale ci consegna ogni giorno episodi di violenza, spesso efferata, compiuta da immigrati entrati clandestinamente in Italia, nemmeno quando già si erano fatti conoscere dalle Forze dell'ordine per i loro comportamenti delinquenziali. Lasciati liberi e impuniti, molti hanno cominciato a girovagare per le nostre strade, a volte superando i confini, vivendo di espedienti e commettendo reati; oppure, peggio, diventando facile preda dell'islamismo radicale e terroristico. Lo stupro di gruppo da parte di sette egiziani ai danni di una povera ragazzina tredicenne di Catania è l'ennesimo, mostruoso, drammatico e intollerabile episodio di una lunga sequela di crimini commessi da chi è sbarcato illegalmente in Italia. Nessun buonismo, nessuna giustificazione o comprensione è possibile o tollerabile verso gli autori, a cui ci auguriamo la legge infligga la pena più dura e severa possibile. È evidente che, quando si parla di immigrazione clandestina, ci sono sempre in gioco la sicurezza delle nostre città, l'ordine pubblico e la coesione sociale e a farne le spese sono - come immaginabile - i cittadini appartenenti ai ceti sociali più umili e indifesi. Penso a quelli italiani, ma anche a quei cittadini stranieri regolari che vivono nelle periferie più difficili delle nostre città e si trovano a combattere contro l'ulteriore e inarrestabile degrado del loro ambiente di vita. È per tutto questo che, nell'esprimere il convinto appoggio della Lega al Protocollo d'intesa tra Italia e Albania, chiediamo al Governo di insistere con coraggio, impegno e determinazione per vincere questa battaglia. Ne va del futuro dell'Italia, della nostra società e dei nostri figli.

di propaganda e cinismo: soldi investiti in un altro Paese, in questo caso l'Albania, in cambio del trattenimento dei migranti. Come a dire: li portiamo lontano, lontano dalle nostre case, dalle nostre paure, dai nostri interrogativi, fuori, in territorio straniero, e il problema è risolto. Tutti sappiamo che non è così, perché siamo di fronte a migrazioni epocali dovute a guerre e a catastrofi ambientali che stanno squassando il pianeta, che spingono milioni di persone in cerca di salvezza e libertà. Ognuno di noi, nelle stesse condizioni, farebbe lo stesso. Dopo il 7 ottobre la situazione è ancora più drammatica, con il Mediterraneo orientale in fiamme, a pochi passi da noi. Di fronte a tutto questo servirebbero testa e cuore, e una *leadership* europea, una strategia comune. Voi invece fate l'opposto: decidete di agire da soli, di fare una misura che è uno *spot*, che riguarderà, secondo i vostri piani, 3.000 migranti a fronte di oltre 160.000 arrivi in Italia nell'ultimo anno, ad un costo economico altissimo e soprattutto, Presidente, ad un prezzo morale insopportabile sulla pelle di essere di esseri umani delocalizzati, deportati, come fossero pacchi o merce o carico residuale, come è stato detto in modo vergognoso. Un baratto a perdere, per tutti. Pensiamo cosa succederebbe se tutti i singoli Stati europei facessero allo stesso modo, anziché costruire un'unica politica si organizzassero ognuno per conto proprio, per deportare in un paese terzo, terzo, lautamente pagato, i migranti che bussano alla nostra porta. Sarebbe la fine dell'idea di Europa, che è innanzitutto stato di diritto, che è innanzitutto l'affermazione del principio assoluto di non discriminazione. Al cuore di tutto questo c'è il diritto di asilo, un diritto sacro voluto dai nostri costituenti come reazione alle persecuzioni e al totalitarismo. Questo trattato è uno sfregio per la nostra civiltà, per il nome Italia che portiamo. È un precedente pericoloso dal punto di vista giuridico e umanitario, indirizzato unicamente al respingimento e non all'accoglienza, come invece come invece dice l'articolo 10 della nostra Costituzione. In questo trattato c'è un'idea di criminalizzazione dei migranti, di criminalizzazione della solidarietà. Un rovesciamento inquietante di quello che noi siamo, dei valori che tengono insieme la nostra Repubblica e la nostra democrazia. Voi prefigurate per migranti che fuggono da guerre e da persecuzioni una detenzione automatica, arbitraria e prolungata, senza possibilità di assistenza legale e senza diritto di difesa, come è stato denunciato dalla commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa. Dite che questo trattato non riguarderà chi è vulnerabile, ma non c'è nessuna garanzia sulle procedure a tutela dei bambini, dei malati e delle donne in gravidanza. Vi chiediamo allora almeno di approvare i nostri emendamenti per proteggere bambini, madri, donne che hanno subito violenza. Sappiamo già però che non lo farete. Voi introducete di fatto dei respingimenti collettivi, impedendo ai migranti messi in salvo da navi italiane, a cui va sempre tutta la nostra riconoscenza, di richiedere asilo nel territorio dove mettono piede, che è l'Italia - perché quelle navi sono territorio italiano - e non l'Albania. Ricordo che l'Albania è un Paese fuori dall'Unione europea e quindi fuori dalla copertura del diritto d'asilo europeo. evidente come ci sia un inganno e l'aggiramento di un diritto che non è dei migranti, ma è un diritto universale! Stravolgete il sistema di soccorso in mare, negando lo sbarco nel primo porto sicuro utile più vicino al naufragio, costringendo ad affrontare giorni di mare in più per arrivare in Albania, dove voi prevedete di costruire, con costi altissimi, nuovi CPR, CPR, nuovi "centri di permanenza per il rimpatrio", come quelli famigerati che ci sono in Italia. Centri dove sono ammassate, spesso in gabbia, in condizioni oltre il disumano, persone che non hanno alcuna colpa, di ventidue anni, che si è tolto la vita a Ponte Galeria, pochi giorni fa, lasciando un messaggio che è un monito durissimo verso la nostra indifferenza. noi chiediamo che questi centri vengano chiusi, in Italia, in Albania, ovunque. Noi chiediamo che le risorse enormi qui stanziate, pari quasi a 700 milioni dei contribuenti italiani, vengano utilizzate per scuola, sanità, lavoro o siano utilizzate per costruire integrazione e inclusione, quel sistema di accoglienza diffuso imperniato sui Comuni e sull'associazionismo laico e religioso, che voi avete smantellato, ma che è invece l'unico che può creare sicurezza per tutti, Presidente, noi voteremo contro questo disegno di legge perché viola quel che di più importante abbiamo, il codice dei diritti, il codice dell'umanità: tutti gli uomini sono creati uguali e, tra i loro diritti, tra i nostri diritti inalienabili, ci sono la vita, la libertà, la felicità. Questi ideali saranno più forti del vostro Governo e noi continueremo a batterci per farli vivere.

degli esponenti dell'opposizione e si sia concretizzato in un legittimo ostruzionismo in Commissione, nonostante il calendario votato all'unità nella Conferenza dei Capigruppo. Siamo qua oggi a discutere questo provvedimento, seppur con diversi giorni di ritardo, rappresenta ai testimoni non solo il fatto che stiamo andando nella giusta direzione, ma anche il fatto che anche sul tema dell'immigrazione siamo ed eravamo pronti. Eravamo pronti sui temi dell'economia. Basta guardare i numeri. Abbiamo il più alto livello di occupazione degli ultimi quarantasei anni, la disoccupazione più bassa degli ultimi diciannove. Eravamo pronti sul tema del contrasto alla povertà, visto che continua ad aumentare, anche se non abbastanza, la capacità per le famiglie italiane del loro potere d'acquisto. Eravamo pronti a invertire la rotta sulla sanità, perché dopo i 37 miliardi di euro tagliati dai Governi della sinistra nel periodo 2012-2018 invertiamo la rotta e abbiamo la più alta spesa sanitaria nella storia repubblicana prevista per l'anno solare in corso. Eravamo pronti sui temi dell'immigrazione, perché i citati decreti messi a sistema col Piano Mattei testimoniano un semplice fatto: il cambio di paradigma nei confronti dei rapporti con i Paesi africani rispetto all'atteggiamento che l'Europa ha avuto negli ultimi duecento anni. Ed è abbastanza singolare, se non bizzarro, il fatto che coloro i quali ci vengono spesso indicati come esempi da seguire in Europa altro non sono che quelle Nazioni che più hanno perpetuato ed agito in modo predatorio nei confronti dei Paesi africani. Noi sosteniamo che il dramma dell'immigrazione, partendo dal concetto già citato del diritto a non emigrare, sia quello che va messo a sistema non solo con un intervento, ovviamente, a difesa delle nostre frontiere, perché i confini sono sacri e come tali vanno difesi, ma con uno sviluppo di quelle Nazioni che hanno la possibilità, nella ricchezza del loro sottosuolo, di trovare risorse per poter crescere e migliorare la loro condizione.

quanto ai rapporti tra Italia e Albania, il primo accordo bilaterale di amicizia risale al 1995 con il Governo Dini, al cui interno era prevista la possibilità di collaborare proprio in tema di immigrazione irregolare; un altro accordo c'è stato nel 2017, sempre con Governo a guida centrosinistra, tra il Ministero dell'interno albanese e il Ministero dell'interno italiano, e ancora una volta si prometteva un reciproco aiuto nel contrasto all'immigrazione. fa altro che concretizzare l'evoluzione di quei passaggi, che questo Stato, non questo Governo, aveva già fatto in passato. Dopodiché, invito gli esponenti dell'opposizione, signor Presidente, a uscire da un provincialismo ideologico che non fa loro onore. Su questa tematica non bisogna ascoltare il sottoscritto o gli altri intervenuti del Gruppo Fratelli d'Italia, o i membri del Governo, ma basterebbe ascoltare cosa hanno dichiarato su questo provvedimento il professor Sabino Cassese, il Presidente emerito della Consulta, il professor Mirabelli, o Pietro Dublino. Signori miei, avete sentito che cosa ha dichiarato il cancelliere socialdemocratico della Germania, Olaf Scholz, su questo, quando i Länder tedeschi chiedevano di guardare al modello italo-albanese rispetto alla possibilità di fare le verifiche per per coloro i quali potessero o meno entrare nel loro territorio, fuori dai confini? Ha detto che guardava a questo accordo con grande interesse, così come ha fatto il commissario europeo per Noi non stiamo vivendo in un contesto - come ci dipingete - lunare, ma forse chi vive sulla luna siete voi, che uscite dai contesti europei in cui un altro paradigma è cambiato, perché l'alternativa ai controlli fuori dai nostri confini nazionali è solo quella della redistribuzione. La redistribuzione è stato dimostrato che non può funzionare, perché sono diversi i Paesi, non solo quelli di Visegrad, che non vogliono accettare gli immigrati che provengono Nazioni. *(Applausi)*. Allora noi comprendiamo - e l'Europa a livello dichiarativo lo sta già facendo - che dobbiamo arrivare a quel concetto geografico e non politico che i confini dell'Italia sono anche i confini dell'Europa e, quindi, chi entra in Italia entra in Europa e che il successivo il successivo passo non può non essere quello di una distribuzione che non funziona. Quella può funzionare ovviamente per i profughi, ma non può funzionare per l'immigrazione cosiddetta irregolare. Allora, l'accordo con l'Albania, al netto delle nefandezze giuridiche che ho sentito, perché la giurisdizione è evidentemente quella italiana e la legge che vige all'interno di questi centri sarà quella italiana, è talmente

tutti gli altri in tema di immigrazione, porteranno l'Italia ad andare in una determinata direzione. Senatore Magni, anche noi non abbiamo la bacchetta magica, non ce l'ha nessuno, ma bisogna capire qual è la direzione in cui si vuole andare: noi l'abbiamo ben chiara e su quella proseguiremo.

Signor Presidente, è doveroso da parte del Governo intervenire su quello che è stato un ampio dibattito, che si è svolto prima alla Camera,

la democrazia ci dà questa possibilità, seppur con visioni completamente differenti. Devo fare una sottolineatura, signor Presidente, tramite la sua persona, ai tanti colleghi che sono intervenuti per quanto riguarda i Gruppi di opposizione. Vorrei dire che spesso il linguaggio in politica è una cosa fondamentale, le parole possono essere pietre e possono destare, per quanto mi riguarda, un po' di stupore. riferisco a chi ha parlato di carro bestiame, a chi ha citato la deportazione, a chi ha parlato di un Governo che si arrende perché non è in grado, perché è impotente. Credo che i veri impotenti siano coloro che non fanno nulla, che non tentano nessun percorso, che si girano dall'altra parte, che si celano dietro l'ipocrisia di una apparente integrazione e di un'apparente accoglienza. Ai quesiti, devo dire molto simili - come è giusto che sia

culturali piuttosto che gli interpreti, rispetto all'assistenza medica e all'assistenza legale; rispetto a un Protocollo che abbiamo messo in campo e che sarà certamente perfettibile, ma che ha delle basi straordinarie per fare quello che il Governo Meloni sin dall'inizio ha

la possibilità di costruirsi un futuro e una storia, di non dividere quelle famiglie che tanto preoccupano qualcuno, e quindi di poterli far rimanere nella propria terra.

marginalità e a ciò che poteva essere visto tanto tempo fa e negli ultimi dieci anni, rispetto alle violenze sulle donne, rispetto ai centri che ho girato in lungo e in largo e che abbiamo trovato in situazioni

Ho sentito dire in qualche intervento che il ministro Piantedosi aveva accennato alle dieci strutture dei CPR. Su questi temi, ovviamente, ci siamo mossi - come è giusto che faccia un Governo - con serietà e affidabilità, attraverso la ricerca di aree apposite che abbiano dei requisiti, attraverso dei sopralluoghi congiunti con il Ministero della difesa e attraverso quelle procedure che dovranno essere messe in atto per realizzare quelle strutture in modo intelligente e soprattutto affinché

senza nessuna forma di strumentalizzazione. Io mi auguro che siano gli italiani a decidere se il nostro *premier* Meloni ha quella credibilità che tutti le riconoscono, ma che soprattutto mi auguro debba essere riconosciuta *in primis* dagli italiani e non da qualche Gruppo che fa parte di questo autorevole Senato.

preparazione e studio. Vorrei dire che l'azione di questo Governo - deve essere chiaro - è e resterà sempre ispirata all'umanità e alla fermezza. Non abbiamo nessuna intenzione di venire meno a quei doveri di accoglienza e di solidarietà verso le persone in fuga da guerre e da persecuzioni; al contempo, però, affermiamo con grande determinazione il principio che in Italia non si entra illegalmente, che la selezione all'ingresso del nostro Paese non sarà fatta dai trafficanti di esseri umani. Vogliamo governare i flussi anziché subirli e vogliamo soprattutto farlo con riforme strutturali, come il Piano Mattei. Bisogna riconoscere senza ipocrisia che l'accoglienza ha certamente un limite invalicabile nella capacità, da parte dello Stato che accoglie, di garantire un'integrazione concreta ed efficace coniugando sicurezza, legalità e coesione sociale, quello che i nostri cittadini ci chiedono. Gli indirizzi del Governo sulle politiche migratorie sono molto chiari e la priorità assoluta è la tutela della dignità della persona. L'Italia conosce bene il significato della parola dignità, anche come parametro di condotta. L'attenzione alla dignità non può fermarsi - come è avvenuto nel corso di tanti anni - alle soglie dei centri di accoglienza. Il dovere dell'Italia è garantire dignità a chi accoglie e a chi è accolto. Non ci sono, purtroppo - ahimè - solo tanti morti in mare, ma anche chi si trova schiavo, costretto nei ghetti ad essere la manovalanza della criminalità, del caporalato, ad essere continuamente sfruttato da chi dell'accoglienza ha fatto una questione di *business.* Credo che la recente sentenza che ha condannato a vent'anni lo scafista di Cutro ne sia un esempio. La solidarietà non può fermarsi, quindi, alla banchina di un porto senza poi garantire quella reale integrazione e la prospettiva di un futuro dignitoso. ci fermiamo a quella giornata, allo sbarco, per poi vedere degli invisibili che camminano sulle nostre strade, di cui ovviamente fino ad oggi nessuno ha avuto cura. Umanità è accogliere i profughi che scappano dalla guerra, dalle persecuzioni, non far scendere migliaia di migranti dai barconi per abbandonarli al proprio destino. Io credo che umanità sia dare finalmente alle persone la scelta di poter decidere di rimanere nella propria terra, di non dover partire per costrizione, lavorando per lo sviluppo dei loro Paesi, anziché sfruttarli con le politiche coloniali. Questo intende fare il Governo Meloni attraverso il Piano Mattei. In vari interventi

al cuore, che è la mano: la mano nel saper decidere, nel sapersi assumere delle responsabilità, come questo Governo sta facendo rispetto a questo Protocollo. Voglio anche ricordare che c'era molto scetticismo per il Protocollo in Tunisia, degli arrivi del 42 per cento. Magari potremo anche sbagliare, ma abbiamo avuto il coraggio di voler fare qualcosa, di non girarci dall'altra parte, di non dare quell'ipocrita accoglienza che ad oggi, purtroppo, non ha dato grandi effetti.

la volontà di far battere le ali e di tentare un futuro diverso, che faccia realmente dell'umanità e della dignità una regola e non un'eccezione. *(Applausi)*.

io ancora non ho avuto risposta, tramite lei, dalla sottosegretario Ferro, che ringrazio per tutto il lavoro fatto in Commissione. Non ho ancora capito quale sia o quali siano le casistiche previste da questo comma 2, che si aggiungono alle operazioni di soccorso in acque internazionali. Al comma 2 si dice che: «nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso». Quali sono le caratteristiche che si aggiungono a questo, per non dover togliere il termine "anche"? Che cosa avete previsto, oltre al salvataggio in mare nelle acque internazionali?

ho voluto prendere la parola su questo emendamento, perché, rispetto a quelli che seguono, esso è particolarmente esplicativo del del nostro intendimento politico e, al tempo stesso, di quanto questo provvedimento sia del tutto irragionevole e privo di qualsiasi giustificazione. Nell'emendamento noi specifichiamo che non possono comunque essere trattenuti nei centri ipotizzati nel territorio albanese le persone che hanno necessità di urgenti cure, le quali potrebbero venire lese nel fondamentale diritto alla salute nell'ulteriore spostamento: minori non accompagnati, donne incinte, ma soprattutto stranieri che hanno titolo per presentare in Italia domanda di protezione internazionale e che, di conseguenza, vengono destinati in un luogo nel quale sarà più difficile per loro esercitare un diritto che la nostra Costituzione e le norme internazionali garantiscono in maniera inequivoca. Ora, respingere questo emendamento disvela tutta l'irrazionalità e l'assurdità di questa misura. Mi spiace non avere il tempo per illustrarlo in maniera più accurata, ma, se i colleghi avranno la pazienza di leggerlo prima di pronunciarsi, credo che farebbero fatica a respingerlo.

l'emendamento in questione è molto delicato, perché parla dei temi legati ai minori non accompagnati, alle donne incinte e alle persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. È bene che si sappia che, così come è stato appurato nel corso dei lavori della Commissione, non è previsto alcun principio di garanzia, tutela e reciprocità fra l'ordinamento della Repubblica italiana e l'ordinamento della Repubblica di Albania. Tradotto: se rimanesse aperto il cancello di questi centri e minori non accompagnati, donne incinte e persone bisognose di cure urgenti ed essenziali uscissero per vari motivi dal cancello di questi CPR, essi rientrerebbero nella competenza piena ed esclusiva della Repubblica di Albania, senza alcuna garanzia in alcun modo assicurata. Credo che questo sia un elemento di grave *vulnus* giuridico, che deve essere oggetto di una modifica. *(Applausi)*. È per questo motivo che noi voteremo a favore di questo emendamento. Chiediamo che l'Assemblea consideri con grande attenzione questi aspetti, che pure dovrebbero essere nel recepimento delle convenzioni internazionali già sottoscritte dal nostro Paese, a tutela di questi soggetti fragili, e che in questo testo legislativo non vengono in alcun modo considerati.

di opposizione. Chiediamo alla maggioranza se cede i propri minuti all'opposizione *(Commenti)*, altrimenti, essendo il tempo contingentato, davvero non riusciamo. senatore Romeo cede parte del suo tempo al senatore Giorgis. Quindi le do due minuti per svolgere la sua dichiarazione di voto. come possono persone che hanno titolo per soggiornare in Italia essere trasferite in luoghi al di fuori del territorio italiano?

G3.102, espungendo le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a favorire la realizzazione di corridoi umanitari per l'ingresso di donne, uomini e bambini profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone».

paragrafo 1, lettera *c)*, a parlamentari italiani ed europei secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia».

espungendo le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a favorire la realizzazione di corridoi umanitari per l'ingresso di donne, uomini e bambini profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone».

da tanti operatori e da tante organizzazioni. Non riesco a capire perché il Governo non possa accettare di avere una relazione semestrale su un'innovazione, su un qualcosa che nessuno ha mai provato prima. Dovrebbe essere interesse di tutti, anche dei parlamentari della maggioranza, ricevere una relazione semestrale per capire come sta funzionando, quali sono le criticità e qual è l'impatto finanziario di questo Protocollo. Mi sembra una cosa di buon senso. nel riconfermare il voto favorevole del Partito Democratico mi appello anche alla maggioranza, perché davvero si tratta di un ordine del giorno di massimo buon senso che garantirebbe ancor più che l'opposizione, la maggioranza rispetto a un Protocollo che oggettivamente ha delle criticità che hanno messo in evidenza tutti e sarebbe garanzia per tutti avere prontamente, ogni sei mesi, una relazione puntuale su ciò che funziona e non funziona di questa sperimentazione.

G4.100 è favorevole, espungendo ovviamente le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare il diritto all'assistenza e alla difesa legale».

Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto favorevole a questo articolo per ringraziare il presidente Balboni che ha dimostrato un grande rispetto dei commissari

Con questa dichiarazione, però, voglio anche ringraziare i colleghi dell'opposizione, perché questa settimana ci è servita per capire bene il senso della norma e gli emendamenti che abbiamo presentato. Pensate che ne abbiamo visti e discussi più di cento, quindi è stato un lavoro utile e propositivo. Per quanto riguarda l'articolo 4, che ci accingiamo ad approvare, volevo solo sottolineare che

ha evidenziato ancora una volta come l'ufficio legale della Commissione europea non ravvisi alcuna violazione del diritto dell'Unione, non essendo lo stesso applicabile al di fuori di essa. Un altro aspetto che riguarda sempre la giurisdizione è quello relativo

Soltanto un piccolo commento: durante la discussione generale mi è capitato di sentire l'intervento di alcuni colleghi di maggioranza ringrazio il collega Liris che mi sta facendo squillare il telefono - i quali hanno detto, restando seri, che Governo e maggioranza lavorano con efficacia e serietà sull'immigrazione, mentre le forze di opposizione fanno soltanto propaganda. Ora, dire che è l'opposizione a fare propaganda sull'immigrazione e non la maggioranza, proprio su questo tema, lo ritengo surreale, perché è stata proprio la propaganda del centrodestra, soprattutto sull'argomento (mi lego alle questioni finanziarie), a creare in questo Paese un profilo di intolleranza nei confronti del fenomeno delle migrazioni. Ricordo sempre i 35 euro al giorno che venivano rinfacciati per la gestione del fenomeno migratorio, come se la dignità umana potesse avere una quantificazione economica in euro.

Era stato aggredito a piazza Gondar, a Roma, mentre attaccava dei manifesti, colpito alla testa da una spranga o da un sasso, non si sa bene da che cosa, perché l'arma del delitto non è mai stata trovata, esattamente come i suoi assassini. Lo vogliamo ricordare perché quella di Paolo è una storia particolare - è al tempo stesso la storia di una generazione, ma anche quella di una nuova idea di destra - ma soprattutto perché con Paolo finiscono gli anni Settanta, esattamente quella mattina, quando con dei lampeggianti blu, insieme a degli agenti di scorta, un Presidente della Repubblica, il partigiano Sandro Pertini, arrivava al Policlinico Umberto I, dove Paolo era in agonia, vegliato dalla sua comunità, i militanti del Fronte della Gioventù. Mentre camminava per quei corridoi, la voce di una ragazza gli disse: Presidente, qui ci ammazzano come cani, perché noi siamo morti di serie B. Il Presidente si avvicinò a quella ragazza e le disse: io sono qui perché voglio condannare chi ha commesso questo fatto esecrabile, da qualunque parte venga. Era la fine di un odioso *slogan* che ci aveva inseguito per tutti gli anni Sessanta e gli anni Settanta, e cioè che uccidere un fascista non era reato, tanto da far scrivere all'allora giornalista di sinistra Giuliano Ferrara su Repubblica: «Abbiamo i titoli per dire che per noi questa non è la morte di un fascista, ma la morte di un uomo. E di più: di dire che se questo scelse di dirsi fascista e concepì per la sua vita futura di vivere da fascista, ebbene, aveva il diritto di scegliere e di vivere così». In realtà Paolo non si era mai definito fascista: come tutta la sua generazione, si riteneva un nazional-popolare, tanto che anche Enrico Berlinguer mandò un telegramma alla sua famiglia, dicendo che era vittima di un'aggressione disumana, che suscitava un commosso compianto anche da parte dei comunisti. Con Paolo finisce un'era, quell'era per cui le famiglie di destra la sera, dopo essersi lavate i denti, prima di andare a letto, mettevano degli stracci bagnati sotto le porte, per evitare di finire come la famiglia Mattei, nel rogo di Primavalle.

Dopo Paolo, quando si tornava a casa la sera, non si faceva più il giro del palazzo tre o quattro volte per paura di un'aggressione; quando si usciva da casa, non ci si fermava più sull'uscio a guardare se c'era qualcuno che aspettava, com'era successo ad Angelo Mancia o a Mario Zicchieri, uscendo da una sezione

Abbiamo vissuto per anni così, semplicemente perché testimoniavamo un'idea. Con Paolo è cambiato tutto, perché Paolo era differente: è morto per attaccare manifesti che volevano restituire Villa Chigi come verde pubblico alla sua comunità di quartiere. Paolo era il capofila di una generazione che si era ribellata al suo partito, perché non voleva raccogliere le firme a favore della pena di morte. Paolo era la teorizzazione della comunità contro la fazione. mentre elaborava le sue idee, i suoi manifesti e le sue teorie, che si doveva riscoprire quella profonda solidarietà e quella nozione di popolo che proprio il predominio della morale mercantile e l'ipertrofia della città avevano distrutto, perché non si fa cultura solo con il libro famoso e con la compagnia teatrale celebre o con il grande film, ma si fa soprattutto con la creazione cosciente del popolo, col suo riunirsi e col suo essere comunità. La nostra nozione di comunità nasce così, anche grazie a Paolo Di Nella. Paolo è stato tutto questo. Paolo era una tenda da campeggio, una motocicletta. Paolo era capelli arruffati e macchie di colla e di vernice sui vestiti.

una promessa, una considerazione e un giuramento: la promessa era che non ci sarebbe stata vendetta, perché per noi gli anni Settanta finivano lì, e che non ci sarebbe stata una scia di sangue che avrebbe coperto altro sangue. Da quel momento in poi, i giovani non si sarebbero più massacrati tra di loro, ma avrebbero scelto solamente idee belle per poter vivere. La considerazione era che non potevamo promettere a Paolo giustizia, perché non dipendeva da noi fare giustizia, era ancora troppo elevata la commistione di una certa magistratura con una certa sinistra, e infatti gli assassini di Paolo e il loro volto non sono ancora noti e non sono stati ancora trovati. Infine, il giuramento: avremmo vinto anche per Paolo. Gli avremmo portato la vittoria come nostro giuramento di una vita politica passata insieme. Io spero che oggi, anche grazie a quello che facciamo, Paolo e i nostri ragazzi lassù sorridano un po' di più.

solamente offrire una testimonianza: ero un po' più piccolo, probabilmente ci siamo incontrati in quei corridoi nell'ospedale.

come tanti altri, ti vesti, prendi il tuo zaino ed esci per andare a scuola, ma c'è qualcosa che ti spinge altrove e ti ritrovi alla stazione a chiedere «scusi, devo prendere il treno per Roma: a che ora passa?». Eh sì, perché a Roma chi c'era mai andato? E poi da solo e per di più con il treno. Ma dovevi andare a vedere come stava quel ragazzo che avevano aggredito a Roma, quel ragazzo chiamato Paolo, che mai avevi visto, ma che sentivi fosse tuo fratello. Un ragazzo che chiamavano rivoluzionario, ma che aveva solo i tuoi stessi sogni, che voleva solo a tutti i costi donare al suo quartiere i giardini di Villa Chigi. Voleva solo vederci giocare i bambini, voleva solo vederci chiacchierare i suoi nonni. Ma per questo fu colpito al capo, forse perché stava dalla parte sbagliata del mondo. Arrivai, non so come, e vidi tanti ragazzi che, a differenza mia, magari ci mia, magari ci avevano parlato e ragionato insieme, che aspettavano in quei corridoi per sapere qualcosa, per sperare di vederlo uscire da quella porta giù in fondo. Eravamo lì ad aspettare Paolo, ma non ci sentivamo assolutamente rivoluzionari, ci sentiamo solamente ragazzi che credevano le stesse cose. Restai lì non so quanto, certamente qualche ora, e poi tornai alla stazione per riprendere quel treno per tornare a Colleferro. Quanti pensieri su quel vagone di ritorno, sperando solo di non essere sgridato dai miei al rientro a casa. Non fu un giorno come gli altri, perché quel giorno segnò profondamente il mio percorso di vita. E se oggi Giorgio è così, tanto dipende anche da quel viaggio in treno e da quell'attesa in quei gelidi corridoi, insieme ad altri giovani "rivoluzionari".

Signor Presidente, ci associamo al dolore, al ricordo e alla ferita perché è una ferita che provoca dolore - ancora aperta per questo anniversario. Mi è capitato altre volte in Parlamento, alla Camera e anche qui, di parlare di quegli anni e di queste cose.

per aprire al pubblico quella villa che era chiusa. A tanti giovani in tutta Italia capitò in quegli anni di fare battaglie anche per aprire spazi di libertà, come il parco di una villa che era chiuso. che era chiuso. Venne sprangato, perché quelli erano gli anni in cui, se uno girava con il «Secolo d'Italia», veniva sprangato. Erano anni in cui, se uno girava con un giornale di sinistra, veniva ammazzato. Per vendetta, alcuni andarono a casa di Valerio Verbano, un ragazzo poco più grande di Paolo, che non era in casa. Suonarono: «Siamo amici di Valerio», dissero ai genitori, che erano lì;

Alla Balduina venne ammazzato Walter Rossi; a Primavalle i fratelli Mattei; a Milano Sergio Ramelli, Fausto e Iaio. Noi abbiamo più volte detto che

a superare quel clima, così come altre manifestazioni di segno opposto non aiutano. Combattiamoci ma, proprio per rispettare questo dolore e per superare quegli anni, evitiamo di tollerare qualsiasi segno estremista che in qualche modo possa far considerare l'avversario ancora oggi un nemico e non un avversario.

Paolo Di Nella, Francesco Cecchin, i ragazzi caduti ad Acca Larenzia, Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti. Non ho conosciuto - perché non si conoscevano ovviamente all'epoca - i caduti dell'altra parte, che pure vanno ricordati, come Walter Rossi e Valerio Verbano, che mi pare di ricordare fu un ragazzo ucciso solo perché stava leggendo «l'Unità» sulla bacheca della sezione del Partito Comunista all'Alberone; trovandosi lì, è morto perché qualcuno ha sparato. Quindi le tragedie sono state molteplici e le ricordiamo tutti. L'amarezza, a decenni di distanza, molte volte è di non aver individuato i colpevoli. Faccio parte di una generazione che nella stessa scuola - ero con Antonio Tajani, che era appena due anni più grande di me Paolo Gentiloni, che era un esponente della sinistra; c'era anche Alvaro Lojacono, che poi abbiamo trovato, secondo le cronache, a Via Fani, con le Brigate Rosse, e che è stato a lungo latitante all'estero, prima di essere assicurato alla giustizia italiana. L'amarezza è per la mancanza di coraggio nell'individuazione dei colpevoli, da un lato e dall'altro. In qualche caso - lo dico al senatore Verini, che questa storia da un altro versante la conosce - ci sono state prove evidenti che sono state ignorate dalla magistratura. Lei, senatore Verini, prima parlava saluti romani ed altre vicende, però su Acca Larenzia la cosa più grave non è tanto chi ha fatto le manifestazioni in un certo modo. Gotor, che è assessore alla cultura al Comune di Roma ed è stato senatore della sinistra, ha scritto un bellissimo articolo su «la Repubblica», ricordando che la parte istituzionale della celebrazione è stata irreprensibile. Poi, ognuno si assuma la responsabilità dei gesti che compie. Stiamo parlando di Paolo Di Nella, che mentre attaccava dei manifesti fu ucciso e morì dopo giorni di agonia. Quella morte, come ha ricordato efficacemente Scurria, segnò una svolta per l'atteggiamento di Pertini - bisogna dirlo - perché le istituzioni per la prima volta ebbero un moto di pietà, che adesso sembrerebbe scontato, ma che allora non lo era (e infatti non c'era stato dopo Acca Larenzia, dopo la morte di Zicchieri e di Mancia), quindi fu il segno di un tempo che per fortuna cambiava. A me dispiace che ancora oggi, a distanza di decenni, non ci siano colpevoli rintracciati in troppe vicende. Si potrebbe parlare di Verbano o di altri omicidi, ma Acca Larenzia la cito perché, più ancora che sulla vicenda di Di Nella, in quel caso è evidente: la mitraglietta che ha ucciso quei ragazzi poi ha ucciso Tarantelli, Lando Conti, Ruffini. Le Brigate Rosse hanno ucciso con la stessa mitraglietta con cui sono stati uccisi Ciavatta e Bigonzetti. Evidentemente, uccisi Ciavatta e Bigonzetti. Evidentemente, alcune persone si sono spostate dai centri sociali della periferia di Roma alle Brigate Rosse, portandosi le armi e nessuno ha fatto un'indagine. Questa è una vergogna che ricade sulla procura della Repubblica di Roma, perché quel reato non è prescritto *(Applausi)* e ci sono libri di giornalisti che descrivono i fatti. nel ricordare Paolo Di Nella, faccio anche un invito dal Senato alla procura di Roma ad indagare. Ci sono elementi e si può fare; sono reati che non si prescrivono su tutte queste vittime. Ho fatto un elenco, che però - ahimè - si potrebbe estendere ulteriormente. In quel caso, che non è quello che ricordiamo oggi di Di Nella, c'è una traccia evidente che è stata ignorata. Siccome ero in una scuola in cui c'era Alvaro Lojacono, che a noi non ha sparato, ma altre persone le ha uccise per strada, vorrei che ci fosse un po' di giustizia per tutti questi caduti. La procura della Repubblica di Roma fa ancora in tempo: ci sono libri di giornalisti, basta consultarli, ce n'è è uno di Nicola Rao molto chiaro ed efficace. Li leggano e facciano quello che è un loro dovere. Noi dobbiamo onorarli con il ricordo, qualcuno potrebbe onorarli colpendo e condannando i colpevoli, nei confronti di tutti coloro che sono morti.

un deputato della VII e della VIII legislatura, poi venne eletto al Senato, sempre nella Democrazia Cristiana, nel 1983 e nel 1987; morì durante la X legislatura da senatore in carica. Bruno Kessler è un personaggio di primissimo piano nella storia della politica del Trentino; è uno di quegli uomini di potere che, per capacità progettuale, *leadership* politica e dinamismo, ha ancora qualcosa da suggerirci a cento anni dalla nascita, perché è stato un uomo di visione, come sottolineò il suo grande amico Beniamino Andreatta durante le esequie nel 1991, ma anche un uomo di granitica convinzione. Questa doppia attitudine bene emerge dalle seguenti parole pronunciate nel lontano 1970: oggi dobbiamo avere il coraggio di inventare, anche sbagliando; dobbiamo avere fierezza e fantasia. Fierezza, cioè crederci capaci di influire sulle cose, nonostante ogni giorno sperimentiamo tutti i limiti dello sforzo compiuto, sia a livello locale sia a livello mondiale. Fantasia, come capacità di anticipare il futuro con coraggio e lungimiranza. I modelli vecchi, collaudati e sicuri, non bastano più. Dobbiamo volere e vedere qualche cosa di nuovo, di duttile, di empirico, oltre le leggi, sopra le leggi, forzando per averne di nuove, che magari lascino ampi spazi a iniziative locali. Kessler nasce il 17 febbraio 1924 a Cogolo di Pejo, un paesino della Val di sole; orfano di padre a quattro anni, la madre lavora ai campi e lui studia in convento per necessità e si laurea in giurisprudenza a Padova. Uomo spigoloso, solitario, politico accentratore, Kessler si iscrive alla DC nel 1945 e diventa segretario di una piccola sezione a ventun anni. Il Trentino dei primi anni Sessanta ha molti problemi e limitate competenze per risolverli da sé; l'aspettativa di vita alla nascita per gli uomini è di sessantadue anni, la più bassa d'Italia; il reddito è al di sotto della media nazionale; si registrano forti tassi di emigrazione e alte punte di disoccupazione stagionale; l'occupazione femminile extradomestica è scarsa, mancano servizi e infrastrutture, soprattutto nelle valli. La parola d'ordine in quegli anni di riformismo politico è ovunque programmazione. Kessler la fa propria ed elabora un progetto organico per la modernizzazione della sua terra, anche attraverso l'investimento in cultura e ricerca. Kessler aveva capito che il riscatto di una terra marginale e povera non passava solo dal miglioramento delle condizioni materiali di vita della popolazione, ma da un più ampio processo di crescita culturale. Assegnava in particolare all'università un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio. Così prende forma l'idea, che poi diventa disegno politico, della prima facoltà di sociologia in Italia. Kessler tocca con mano una scienza nuova, almeno in Italia: la sociologia. In questa disciplina, dotata di strumenti empirici duttili per leggere quel presente complesso, Kessler vede un futuro, ovvero la possibilità di formare una classe dirigente all'altezza dei tempi nuovi, di favorire la sprovincializzazione del Trentino. Così nel 1962, per ovviare all'impossibilità giuridica della Provincia di fondare direttamente un istituto universitario, nasce l'Istituto trentino di cultura. Kessler dovrà affrontare diversi ostacoli per veder compiutamente realizzato il suo progetto. Sociologia sarà la prima università di massa, nel senso che è la prima ad aprire le porte anche ai diplomati degli istituti tecnici. Egli non è solo: lo aiutano innanzitutto padre Luigi Rosa dei Gesuiti di San Fedele a Milano e studiosi come Marcello Boldrini, Giorgio Braga, Mario Volpato, l'amico Beniamino Andreatta e poi Norberto Bobbio, Paolo Sylos Labini, Alessandro Pizzorno, fino a Francesco Alberoni. Trento, capitale della sociologia, è però solo il primo frutto del modello autonomistico kessleriano, la nascita di nuove facoltà e la creazione di istituti di ricerca di alto profilo scientifico e internazionale. Vengono fondati nel 1973 l'Istituto storico italo-germanico, nel 1975 l'Istituto di scienze religiose e nel 1976 il Centro per la ricerca scientifica e tecnologica, nato come Centro di sviluppo e ricerca in fisica, che sarà uno dei primi centri in Italia a occuparsi di intelligenza artificiale con il professor Luigi Stringa. Concludo dicendo che il Trentino doveva appropriarsi in modo più convinto della propria autonomia, ancorandosi alla solidità delle proprie tradizioni non come a una zavorra, ma come a una spinta verso l'apertura e l'innovazione. Questa è l'idea che sta alla base dell'originale progetto di Bruno Kessler: una comunità che trova riscatto nella conoscenza e cresce nel sapere dovrebbe essere ancora il punto da cui partire per rinnovare il tessuto economico, sociale e culturale di un territorio. Desidero, in conclusione, ringraziare soprattutto la figlia Elisabetta Kessler, che appunto ieri era qui con noi e anche Sara Zanatta, sociologa di quella facoltà aperta grazie a Bruno Kessler, attualmente ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino che ha collaborato con me per la ricostruzione di questi aspetti. *(Applausi)*.

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, lo scorso 9 febbraio è stato il terzo anniversario della morte del Presidente emerito del Senato Franco Marini. Egli ha quest'Aula con autorevolezza e spirito costituzionale, come è stato per tutta la sua vita e nei molti ruoli di servizio al Paese. Franco Marini è stato capace di coniugare in sé l'uomo di parte, con la sua passione autentica, e l'uomo delle istituzioni, sempre capace di più avanzate mediazioni per il bene comune. Ha sempre ricercato l'unità e lavorato per essa nel partito, come nei ruoli che ha ricoperto, guardando agli ultimi e all'equità sociale come obiettivo prioritario del suo servizio. Equità, giustizia sociale, dignità del lavoro: una ragione di vita fatta propria sin dalla più giovane età, quando il "lupo marsicano" girava la Marsica in bicicletta per raggiungere i luoghi di lavoro e di lotta sindacale. Da lì fino alla segreteria generale della CISL, poi le istituzioni: da Ministro del lavoro, darà alla luce la legge n. 460 del 1992, una normativa dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici con l'introduzione di ammortizzatori sociali e sostegno all'occupazione; ne era orgogliosissimo e non perdeva occasione di ricordarlo. Ma furono quelli anche gli anni di collaborazione con Mino Martinazzoli come capo dell'organizzazione nazionale della Democrazia Cristiana, un ruolo che poi lo porterà nel 1997 alla segreteria del Partito popolare italiano. Marini ha attraversato quegli anni da assoluto protagonista, *leader* riconosciuto, spesso decisivo nei principali snodi politici. È stato uno dei padri della coalizione di centrosinistra, dalla nascita della Margherita alla fondazione del Partito Democratico, del quale è rimasto, fino alla fine, un forte punto di riferimento. Una vita da combattente, da uomo delle istituzioni. Credeva nei partiti, nella militanza, nell'impegno nella partecipazione, nella politica popolare in grado di stare fra le persone, in grado di farsi capire sempre dalle persone. Sarebbe stato un grande Presidente del Consiglio, in quel 2008 in cui il presidente Napolitano gli affidò il mandato esplorativo, e sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica. In quest'Aula ci sono voci molto più autorevoli della mia che potrebbero ricordare meglio una vita politica così lunga e intensa: il senatore Dario Franceschini, il più importante allievo, figlio politico e amico, la senatrice Annamaria Furlan che parlerà dopo di me, prima donna segretaria generale della CISL, chi era in Senato durante la sua Presidenza, chi ha collaborato gomito a gomito con lui nel Partito Nazionale. Io, di quarantacinque anni più giovane, ho solo due piccole ragioni per parlare qui ora. La prima è la condivisione delle comuni radici abruzzesi; la seconda è la fortuna di aver avuto il suo severo affetto nei miei primi impegni politici territoriali. La sua postura, la chiarezza, la lucidità, la ruvidezza coriacea, il richiamo costante e fermissimo alla realtà dei fatti, la giovialità nei convivi, accompagnati dai canti degli alpini, la direzione, condotta non come il generale chiuso nella sua tenda nelle retrovie, ma davanti, a segnare il passo: non aveva niente della pedanteria professorale, ma era comunque un grande maestro, nel solo modo in cui in politica forse lo si può essere, ossia con l'esempio. Questo mio, allora, vuole essere solo un abbraccio al figlio Davide ed un monito a noi. Franco Marini merita molto di più di tre minuti, non solo per lui, ma per noi, per le istituzioni, per il dialogo fra le parti sociali, per la comunità nazionale, per il futuro del nostro Paese.

Mi fa effetto parlare di Franco Marini in un'Aula semivuota, che avrebbe, per la caratura morale, etica della persona, per il ruolo istituzionale e sociale, meritato una presenza molto più numerosa. Ma avremo - io spero - altre occasioni. Io ringrazio di cuore le amiche e gli amici della maggioranza e dell'opposizione che hanno voluto fermarsi e condividere con me e il senatore Fina queste due riflessioni. Franco è stato per me, come per tanti della mia generazione della CISL, un grande maestro:

vita è stato rivolto agli ultimi, alla tutela dei più deboli e alla centralità del ruolo sociale del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Con questo spirito egli è stato un grande segretario generale della CISL. Ha saputo costruire momenti di unità sindacale molto forti, tenendo sempre però fermi quelli che sono stati i principi di libertà, di eguaglianza, di democrazia che hanno caratterizzato la vita della nostra organizzazione e la nascita della CISL. Con questo spirito ha portato, nelle istituzioni e nel suo percorso politico, il valore sociale della persona nel lavoro. Non c'è stato un attimo, nemmeno un secondo, anche della sua attività istituzionale e politica, in cui non abbia sempre messo al centro il lavoro come elemento di crescita della persona, di una comunità, di un partito, ma anche di un Paese. A lui dobbiamo tantissimo. Alle volte qualcuno mi ha chiesto: dove è andata l'eredità morale e politica di Franco Marini? Credo che non esista una sola persona, nemmeno un solo partito, così profondi da poter ereditare da soli l'esempio di Franco Marini. Sono le istituzioni che ricevono, dai grandi uomini dalle grandi donne che hanno dedicato una vita alla democrazia e al Paese, la loro eredità morale, etica e di esempio. ringrazio per avermi dato la parola. Io ho ascoltato con attenzione e con emozione quanto hanno detto il senatore Fina e la senatrice Furlan. mi associo a tutto quello che i colleghi hanno detto, pur da parte politica diversa. Io vissi quella legislatura che vide il presidente Marini Marini rivestire la seconda carica dello Stato, come Presidente del Senato. Fu una legislatura turbolenta fin dall'inizio, fin dall'elezione stessa di Franco Marini, che fu disputata e fu all'ultimo voto. Ma il presidente Marini seppe conquistarsi la fiducia e il rispetto di tutte le parti politiche, pur avendo appunto un compito estremamente difficile, per quel lato umano di cui avete parlato. Non aggiungo altro, perché chi l'ha conosciuto meglio e chi gli è stato più vicino più vicino ha titolo per dire di più. Il suo lato umano, la sua sensibilità politica, l'agire non per un ideale astratto, ma per le persone, nell'ambito di un ideale, di un pensiero e di una cultura, credo siano stati il tratto caratterizzante di Franco Marini e di tutti quelli che hanno avuto l'onore e il piacere di incontrarlo e di avere avuto momenti di amicizia con lui. A nome A nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, mi associo a questa commemorazione, che è commovente e ricorda pagine importanti di questa istituzione. finestra"). La Presidenza si associa al ricordo del presidente Marini e alla vicinanza espressa alla sua famiglia. Ci tengo a dire che questa non era una commemorazione programmata, per cui i colleghi chiaramente non erano informati del contenuto degli interventi